sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*. Invito i senatori Segretari a

del 16 marzo 2006 (reato transnazionale)». La richiesta è stata trasmessa dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma il 20 giugno 2022. La relazione è stata stampata e distribuita. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per tutte le imputazioni contestate, attesa la sussistenza nel caso di specie dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1

Signor Presidente, anche se lei ha già anticipato gran parte del contenuto, credo possa essere opportuno ricordare ai colleghi l'accaduto, l'attività della Giunta e, seppur brevemente, il tema che stiamo trattando. Come lei ha anticipato, in data 20 giugno 2022, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, in conformità a quanto disposto dal Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma, con relazione depositata il 16 giugno del 2022, ha trasmesso al Presidente del Senato della Repubblica gli atti del procedimento penale, sezione reati ministeriali, nei confronti del dottor Corrado Clini, nella qualità di ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore*, per l'avvio della procedura di cui all'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989, ai fini del rilascio dell'autorizzazione in ordine ai reati di cui agli articoli 416 del codice penale (associazione a delinquere); 81 capoverso, 319 e 319-*bis* del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio continuata e aggravata), 110 e 353 del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); con l'aggravante di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 146 del 16 marzo del 2006. La complessa vicenda, colleghi, contestata all'ex ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dottor Corrado Clini, è stata poi illustrata nella seduta della Giunta del 7 marzo 2023, al cui resoconto si rinvia.

Dicevo che preliminarmente si precisa sul piano metodologico che l'autorizzazione a procedere di quel combinato disposto dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del applicabile ai soli reati ministeriali, ossia per i reati commessi dal ministro in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, differisce totalmente dall'inviolabilità prevista al secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione. L'articolo 9, comma 3, della citata legge costituzionale delimita espressamente l'oggetto della valutazione del Senato, richiedendo che quest'ultimo focalizzi la propria istruttoria esclusivamente su due circostanze distinte tra di loro, ossia sul fatto che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il proseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, congiuntamente al preliminare accertamento circa la natura ministeriale del reato che ad essa è strumentale. La prima decisione, quindi, che la Giunta è stata chiamata ad assumere è quella attinente alla verifica della sussistenza della natura ministeriale del reato, che si configura quindi come una precondizione necessaria, ma non sufficiente. Un reato può essere infatti valutato come ministeriale in quanto commesso in occasione dell'esercizio di funzioni ministeriali e, tuttavia, non essere ispirato dalle finalità di tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. Si evidenzia che il tribunale dei Ministri ha ravvisato la natura ministeriale ed ha conseguentemente rivolto al Senato l'autorizzazione a procedere per tale tipologia di reati. Si ritiene che tale tesi sia condivisibile, atteso che nel caso di specie è sicuramente ravvisabile la ministerialità del reato, dal momento che tutti i fatti dei quali è accusato il dottor Clini sono riconducibili alla competenza funzionale dello stesso quando era in carica come Ministro. La Giunta è stata inoltre chiamata a verificare, in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, in merito alla sussistenza di una delle due scriminanti previste dal citato articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, e cioè se il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. L'inciso: «con valutazione insindacabile» contenuto nella disposizione costituzionale in questione costituisce un *unicum* nell'ambito della normativa di rango costituzionale, nel senso che in nessun'altra disposizione si precisa che la valutazione della Camera competente è insindacabile. Tale circostanza conferma ulteriormente l'attenzione che ha posto il legislatore costituzionale all'autonomia del Parlamento, precludendo alla Consulta un sindacato di merito sulle valutazioni su tale scriminante *extra ordinem* effettuate dalla Camera competente. Nel caso in esame non appare configurabile la prima delle esimenti previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989; mentre si può ritenere che ricorra la seconda delle scriminanti in questione, ossia quella del perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo. È necessario precisare che, per il diniego dell'autorizzazione a procedere, il comma 3 sopra citato richiede la ricorrenza di una o dell'altra scriminante alternativamente e non quindi cumulativamente, come evidenziato dalla locuzione «ovvero». Con riferimento alla seconda delle citate scriminanti, occorre chiarire che un Ministro potrebbe anche aver perseguito un preminente interesse pubblico, senza però che tale sua finalità possa essere riconducibile all'esercizio della funzione di Governo. La legge costituzionale non cita l'esercizio della funzione di Governo casualmente, ma lo fa con un obiettivo specifico, ossia quello di garantire la salvaguardia dell'autonomia di tale funzione nei casi in cui la stessa sia rivolta al perseguimento di un preminente interesse pubblico. Se nella prima scriminante il legislatore parla di interesse dello Stato, nella seconda fa riferimento al preminente interesse pubblico, concetto non coincidente del tutto con il primo. Inoltre, nella prima scriminante si dice che il Ministro deve avere agito per la tutela di un interesse dello Stato, mentre nella seconda si parla di perseguimento di un preminente interesse pubblico e non quindi di tutela di tale interesse, in modo tale da valorizzare il profilo teleologico della condotta del Ministro. al caso di specie, la condotta del ministro Clini relativamente al Montenegro si colloca in un contesto politico istituzionale piuttosto ampio, senza ombra di dubbio riconducibile all'azione di Governo. Occorre a tale proposito rammentare che l'allora presidente del Consiglio Monti, nell'esporre il programma di Governo dinanzi al Senato della Repubblica il 17 novembre 2011, richiamava da un lato - il risanamento della finanza pubblica e il rilancio della crescita, che avrebbero dovuto contribuire a rafforzare la posizione dell'Italia in Europa e più in generale la nostra politica estera; dall'altro, la vocazione europeistica del nostro Paese, sottolineando peraltro come l'Italia abbia bisogno di una politica estera coerente con i nostri impegni e di una ripresa di iniziativa nelle aree dove vi siano significativi interessi nazionali. A tali dichiarazioni programmatiche facevano peraltro seguito, in data 22 novembre 2011, le comunicazioni del dottor Clini in qualità di Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

nell'esercizio dell'azione di Governo, e in particolare l'interesse pubblico alla cooperazione internazionale in materia ambientale, emerge *ictu oculi* da diversi elementi. A tal proposito si evidenzia che a livello internazionale nel dicembre 2011 il dottor Clini ha guidato la negoziazione italiana nel citato *summit* ONU del clima a Durban, in Sudafrica, e nel gennaio dell'anno successivo ha presentato le iniziative per il Vertice mondiale della terra in programma a Rio de Janeiro per il mese di giugno. Nella memoria che il dottor Clini ci ha sottoposto, egli evidenzia come la cooperazione ambientale con Serbia e Montenegro avesse preso avvio già anteriormente alla sua assunzione della carica di Ministro e precisamente da un accordo firmato a Johannesburg nel 2002 dai Ministri dell'Italia e della Serbia in occasione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. In particolare, poi, dopo l'indipendenza del Montenegro nel 2006, il programma di cooperazione ha avuto un ulteriore impulso di espansione, con il supporto del Ministero degli affari esteri e dell'ambasciata italiana in Montenegro. Il dottor Clini ha sostenuto che, in relazione ai progetti sopra citati, la situazione si è posta nel senso di dare attuazione a indirizzi strategici della politica estera italiana e tale affermazione, colleghi, appare suffragata da tutti questi elementi. quanto esposto, come le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i princìpi ispiratori della politica governativa dell'epoca, con particolare riguardo alla vocazione europeista dell'Italia e alle politiche per lo sviluppo e la crescita, trasfondendole nel settore di pertinenza del Ministero dell'ambiente. In questo caso, appare evidente dagli elementi richiamati come il perseguimento di un preminente interesse pubblico sia consistito - da un lato - nel tentativo di promuovere la conversione verde soprattutto dei Paesi di nuova economia e di crescita, tra i quali rientra il Montenegro e - dall'altro - nel promuovere progetti tesi a sostenere l'adesione del Paese balcanico all'Unione europea. conclusione, signor Presidente, la Giunta, per i motivi fin qui evidenziati, propone - come lei ha già detto - a maggioranza all'Assemblea il diniego della richiesta di autorizzazione a procedere per tutte le imputazioni contestate, attesa la sussistenza, in questo caso, dell'esimente del perseguimento del preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989. **Saluto

in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori, che hanno l'occasione di assistere a una discussione su un punto dirimente di applicazione della nostra Carta costituzionale.

elementi che lo rendono molto particolare. Il primo elemento è che stiamo parlando di fatti accaduti tantissimo tempo fa, nel senso che il dottor Clini è stato Ministro dell'ambiente nel Governo Monti,

Il secondo elemento caratterizzante è che in questa vicenda il dottor Clini è imputato per gli stessi fatti sia come direttore generale del Ministero, sia poi a seguire, in una seconda fase, come Ministro dell'ambiente. Quindi, abbiamo due procedimenti che stanno comunque procedendo parallelamente perché il dottor Clini è chiamato a rispondere esattamente delle medesime condotte anche come direttore generale e, in quanto non Ministro, certamente dovrà essere giudicato per quei fatti ed eventualmente sanzionato, sempre che non intervenga la prescrizione perché stiamo parlando di fatti molto antichi. Noi voteremo a favore delle conclusioni Giunta, la complessità della questione rende difficile un giudizio così netto. E spiego anche qual è, dal punto di vista tecnico, la difficoltà che - devo dirlo ai colleghi - anche il relatore, il collega Paroli, durante i lavori ha dovuto evidenziare. C'è stato un momento del nostro lavoro nel quale abbiamo pensato di chiudere per alcuni dei fatti contestati con una certa deliberazione e rimandare gli atti al giudice remittente per altri fatti. In realtà, tecnicamente questo non sarà possibile e, quindi, siamo costretti ad arrivare ad una decisione unica su fatti che però hanno caratteristiche diverse. È diverse. È chiaro che, per esempio, pensare a un reato ministeriale con una turbativa d'asta è più semplice: ammettiamo che nel perseguimento dell'interesse pubblico si siano eccessivamente semplificate le norme procedurali per quell'asta. È chiaro che il Ministro può dire che stava cercando di implementare l'interesse pubblico che, in questo caso, secondo me è fuori discussione, perché la perché la collaborazione con Serbia e Montenegro e in genere con i Balcani occidentali è un elemento caratterizzante della politica estera di tutti i Governi della Repubblica. Per noi i Balcani occidentali sono un luogo un luogo centrale della nostra attività di politica estera, e che il Ministro degli affari esteri facesse di tutto per migliorare e stringere la collaborazione tra il nostro Paese, la Serbia e il Montenegro è assolutamente fuori discussione. Voglio ricordare, per esempio, che non molti anni fa abbiamo steso un cavo per il passaggio dell'alta tensione tra Montenegro e Italia ed è stato un momento molto importante della nostra collaborazione proprio dal punto di vista energetico. Quindi, da questo punto di vista, non ho alcuna perplessità. È chiaro che, quando il giudice remittente costruisce un reato come quello della corruzione, diventa un po' più complicato capire come un fatto di quel genere possa realizzare un interesse pubblico. Devo dire, però, che costretti a decidere nell'interezza; considerato che è fuori discussione il fatto che lavorare con Serbia e Montenegro sia parte della nostra politica estera e della nostra politica energetica e tenuto conto ed è per me l'elemento prevalente - che qualsiasi decisione prenderà l'Assemblea, comunque per quei fatti il ministro Clini sarà chiamato a rispondere in quanto direttore generale. Nella complessità di tutti gli elementi, la nostra valutazione, per non dare un giudizio di astensione - secondo me in casi come questi non è mai appropriato perché, se il giudice richiede un parere richiede un parere vincolante così importante, è giusto rispondere sì o no e lavarsene le mani non mi sembra la soluzione migliore - a nome del mio Gruppo io ritengo prevalenti gli elementi per votare a favore della relazione del collega Paroli. E si vota nella consapevolezza che su quei fatti il giudice ordinario continuerà le sue valutazioni e sarà il giudice ordinario a decidere

Andiamo con ordine: ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Sul punto la relazione proposta è esaustiva e spiega bene cosa si intende per la prima ipotesi, per la seconda; il motivo secondo il quale la fattispecie non ricade nella prima ipotesi è il perché, invece, la condotta dell'ex Ministro potrebbe ricadere nella seconda, cioè per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Tuttavia, a nostro avviso, una valutazione a monte andrebbe fatta. La tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante rappresenta un fine di per sé preminente, volto ad assicurare la sopravvivenza stessa dello Stato, andrebbe inteso quale interesse e presupposto di tutti gli altri interessi. Per quanto concerne invece il perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo, al fine di creare i presupposti per l'applicazione o no della scriminante, andrebbe compiuta una necessaria valutazione di preminenza dell'interesse pubblico rispetto alla confliggente fattispecie incriminatrice oggetto di valutazione; elemento che, per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, non è richiesto. Dalla lettura della relazione conclusiva non traspare alcuna condotta integratrice di reato posto in essere dall'allora ministro Clini, quasi che le ben 34 pagine trasmesse alla Presidenza del Senato dalla procura della Repubblica di Roma, con le quali venivano contestate molteplici condotte di reato all'ex Ministro, non fossero mai esistite. Di conseguenza, a nostro avviso, non è stata compiuta una necessaria valutazione di preminenza dell'interesse pubblico rispetto alle ipotesi di reato contestate. Dalla valutazione della relazione, infatti, appare che la Giunta si sia soffermata solo e soltanto alla mera rispondenza della condotta del Ministro a un interesse pubblico e che tale azione sia in linea con l'esercizio della funzione di Governo. Non si pongono in stretta correlazione le fattispecie di reato con l'interesse pubblico, bensì si mettono in risalto le condotte astrattamente poste in essere dal Ministro con la rispondenza a un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Nella relazione si fa riferimento - cito testualmente - al fatto che «le attività del ministro Clini si pongano in senso coerente con quelli che erano i princìpi ispiratori della politica governativa dell'epoca», ma non si procede a un bilanciamento tra tali politiche e il fatto che il perseguimento delle stesse sia avvenuto mediante condotte atte a integrare i delitti di cui agli articoli 416, 319 e 319-*bis* del codice penale. A questo punto, avendo escluso l'applicabilità della prima scriminante e ricadendo nella seconda ipotesi, la proposta conclusiva del relatore avrebbe dovuto contenere questo giudizio di preminenza; cosa che purtroppo non appare. Si sarebbe dovuta infatti accertare la funzionalizzazione della condotta criminale all'interesse pubblico quindi, che l'associazione a delinquere fosse funzionale al perseguimento del preminente interesse pubblico, ponendosi come unica condotta attraverso la quale perseguire l'interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo, che altrimenti sarebbe stato pregiudicato. Sarebbe stato infatti opportuno che la Giunta, in sede di votazione, avesse valutato le condotte del Ministro anche relativamente ai copiosi investimenti di diversi milioni di euro, presi presi dalle tasche degli italiani, su progetti che intervenivano per abbassare le emissioni in territorio nazionale, aiutando però altri Paesi a ridurre le loro. A me sarebbe piaciuto avere spiegazioni e capire la *ratio*, che mi risulta incomprensibile, di stanziare centinaia di milioni di euro per aiutare un Paese come la Cina, seconda potenza mondiale per il PIL, a disinquinarsi. Nel caso di specie non si riscontra dunque alcun perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo. Si registra piuttosto, come sostenuto tra l'altro dagli organi inquirenti, un interesse privato - questo sì - preminente rispetto al coincidente, ma subordinato all'interesse pubblico. Questo per quanto ottiene al merito. Passiamo al metodo. Neanche la stessa maggioranza è convinta del testo da essa proposto. Ciò si evince anche dallo svolgimento dei lavori che abbiamo avuto in Giunta; in un primo momento era stata formulata una proposta conclusiva, invece oggi ne vagliamo un'altra totalmente diversa, che ha sostituito la precedente. Le due differiscono in maniera sostanziale nel dispositivo. In parole povere e in breve, nella prima relazione conclusiva la maggioranza proponeva una reiezione meramente procedurale invece invece che il rinvio degli atti all'autorità giudiziaria. La prassi consolidata vuole però che, nei casi in cui la Giunta ravvisi l'incompletezza delle indagini, al fine di pervenire a una compiuta valutazione, la stessa richieda di norma il rinvio degli atti. Infatti, siccome l'accertamento del perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio di una funzione di Governo è di competenza della Giunta e dell'Aula, il compito del Senato è formulare questa valutazione politica, non spettando di inquadrarne il profilo giuridico e giudiziario. Relativamente al caso di specie, dunque, non avrebbe avuto formalmente gli elementi per poter decidere sulla questione; quindi la formula della reiezione solo procedurale non sarebbe stata né giustificata, né sufficiente. Forse la maggioranza si è accorta dell'errore e ha stravolto il dispositivo nella seconda relazione conclusiva, che oggi stiamo votando qui in Aula. Ma a questo punto mi chiedo: quali sono gli elementi aggiuntivi che hanno portato la maggioranza a stravolgere la relazione conclusiva, senza che che tra l'altro sia stato trasmesso alcun atto alla Giunta o un ulteriore documento da far cambiare idea al relatore? Altre due valutazioni, se posso, Presidente, desidero svolgere. ordine generale. A nostro avviso, c'è un totale sviamento rispetto al ruolo che il Regolamento del Senato impone alla Giunta. Da organo paragiurisdizionale, che assume decisioni basate su precisi presupposti di fatto e di diritto, si è passati a uno assolutamente politico; anzi in questa circostanza direi politico per eccellenza, che giudica sulla base della forza data dai numeri data dai numeri parlamentari, prendendo quindi decisioni fondate più su presupposti corporativistici piuttosto che su di un attento studio delle carte. A nostro avviso, a questa deriva dobbiamo porre rimedio. E faccio un appello a lei, Presidente. La seconda, più che una valutazione, sono domande che vorrei rivolgere soprattutto ai colleghi della maggioranza. Perché la proposta non è stata votata stessa seduta in cui è stata votata la proposta di Gasparri? Erano insieme nell'ordine del giorno. Perché è stata messa proprio oggi all'ordine del giorno? Perché è stata calendarizzata insieme a un atto che, ai fini dell'approvazione, necessita della maggioranza assoluta dei componenti del Senato? Vi chiedo, colleghi, qual è il *quorum* deliberativo richiesto per le domande di autorizzazione a procedere *ex* articolo 96 della Costituzione? Io ovviamente una risposta me la sono data e non credo che si discosti molto da quella che si daranno i colleghi della maggioranza. Per le ragioni illustrate, sia sotto il profilo del merito che del metodo, e per l'estrema gravità dei reati contestati, esprimo il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

colleghi, l'Aula è piuttosto disattenta, nonostante stiamo discutendo, al di là del caso concreto, un caso

non hanno assolutamente precedenti. Un precedente in termini, quello del ministro Matteoli, era stato giudicato esattamente nel senso di non ritenere

il tenore delle imputazioni per sottolineare, in un clima etico, la gravità delle contestazioni. Il problema non è la gravità delle contestazioni, e cioè corruzione, associazione a delinquere, turbativa d'asta e quant'altro. La questione è che, con queste contestazioni, si contestano delle condotte concrete che hanno al centro un dare e un avere.

un fraseggiare di rito dire che se ne deve occupare la magistratura. Dire, però, che se ne deve occupare la magistratura vuol dire esattamente questo. Qual è il fulcro della nostra decisione? La nostra decisione sta nel fatto che i Padri costituenti hanno stabilito che, qualora ci sia la ragion di Stato al massimo livello, cioè il preminente interesse pubblico, quindi -

come hanno esposto i colleghi che mi hanno preceduto. E io sono veramente incuriosita di come possa reggere, sotto il profilo logico, questa argomentazione. Noi non stiamo discutendo dei rapporti

ad operare dei casi senza precedenti, che travolgono il dettato costituzionale. Noi staremmo per stabilire che, quando c'è un dare e un avere, può essere nell'interesse pubblico. Io vorrei che quest'Assemblea si rendesse conto di che cosa stiamo discutendo. Quando noi abbiamo discusso, per ben tre volte, del caso del ministro Salvini, esattamente sulla sussistenza o meno della scriminante di cui all'articolo 96, naturalmente ci siamo confrontati. Abbiamo votato in modo diverso, giudicando se la condotta,

in una condotta di direzione politica. In quel caso, potevamo pensare diversamente, ma i presupposti per discutere c'erano. Qui, noi stiamo discutendo di un qualcosa per cui mancano totalmente i presupposti

Noi, però, non possiamo entrare nel merito di questi fatti: e non per una eleganza di linguaggio o per un garbo istituzionale. Noi non possiamo entrare nel merito di questo, perché travolgeremmo

fare alcune considerazioni riassuntive, la Giunta non è chiamata a pronunciarsi sulla fondatezza delle accuse. La Giunta prima e l'Assemblea poi hanno solo la possibilità di negare l'autorizzazione a procedere, ove risulti che il Ministro abbia agito a tutela di un interesse nazionale ovvero nel perseguimento di un preminente interesse pubblico. Quelle condotte concrete, però, non si possono cancellare. Il relatore ha provato a cancellarle, in una iniziale proposta di relazione in Giunta, perché era evidente che rappresentavano un ostacolo insuperabile, ma non possono essere cancellate. Noi non possiamo assolutamente giudicare ed acquisire che, se c'è un dare ed un avere, questo dare ed avere può avere la direzione di un interesse pubblico. E vorrei ancora sottolineare che questa scriminante, che deroga alla giurisdizione, è eccezionale. Tanto è vero che le Camere possono negare l'autorizzazione o concederla, ma non si sostituiscono mai alla valutazione del giudice, né possono farlo.

In conclusione, vorrei ancora una volta sottolineare che, tutte le volte che operiamo una torsione che lega le garanzie fondamentali della Costituzione al consenso maggioritario, noi non stiamo affermando il primato della politica. È una discussione di questi ultimi giorni: a me preoccupa molto una sorta di collettiva perdita della cultura costituzionale, che dovrebbe essere assolutamente comune a tutti noi, qualsiasi schieramento politico apparteniamo. Noi travolgiamo i princìpi fondamentali, stabiliti nella Costituzione, del rapporto tra il potere e la libertà dei singoli cittadini, tutte le volte che facciamo prevalere il principio del consenso maggioritario. Non stiamo parlando della ragion di Stato o della ragion di Costituzione, per essere più eleganti con Leopoldo Elia, che non solo è un elegante presupposto e un elegante principio, ma sta anche alla base delle democrazie liberali.

mi stupisco anche del cambiamento di valutazione di alcuni componenti della Giunta, perché il salvagente della complessa imputazione, per cui comunque un giudice si pronuncerà sull'altro aspetto, è assolutamente bucato e non regge il vaglio dell'impostazione costituzionale. Per queste ragioni, voteremo contro le conclusioni della relazione.

del Regolamento, si intenderà respinta qualora non consegua il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Ricordo altresì che il risultato non verrà proclamato immediatamente. I senatori che non abbiano partecipato al voto potranno successivamente recarsi al banco della Presidenza e dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari che ne terranno nota in appositi verbali custoditi. Tale facoltà potrà essere esercitata nel corso della seduta odierna fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista al termine della discussione congiunta della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e della annessa relazione sullo scostamento. Ai sensi dell'articolo 135-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*. I senatori favorevoli alla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere voteranno sì. I senatori contrari alla proposta della Giunta voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

Dichiaro chiusa la votazione nominale con scrutinio simultaneo. I senatori che non abbiano partecipato alla votazione potranno dichiarare il proprio voto palese ai senatori Segretari presso il banco della Presidenza. Tale facoltà potrà essere esercitata fino alla chiusura delle operazioni di voto, prevista al termine della discussione congiunta della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 e della annessa relazione sullo scostamento. termine della discussione congiunta della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023

ci preme precisare e sottoporre all'attenzione della Presidenza, a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico immaginando di interpretare, da questo punto di vista, anche la sensibilità degli altri Gruppi, che la Commissione affari europei non ha potuto esprimere il parere sulla Nota d'aggiornamento al DEF. Non sfuggirà a nessuno dei colleghi non solo l'importanza delle politiche europee, in particolar modo del PNRR su questa Nota di aggiornamento al DEF, visto che due terzi dei risultati che il Governo dice di ottenere nel 2024 dipendono dal PNRR, che è assolutamente inaccettabile che una Commissione così importante non sia stata messa nella condizione di esprimere il parere sulla Nota di aggiornamento al DEF. Sappiamo bene e non è una giustificazione perché non può esserlo, voglio dirlo anticipatamente in relazione ad alcune interpretazioni "larghe" che vengono fatte - che in passato è accaduto che qualche Commissione abbia espresso *ex post* il parere. Premetto che riteniamo questo non corretto, perché la Commissione di merito aspetta i pareri delle altre Commissioni, che sono il risultato di un confronto che è avvenuto, e sulla base di quei pareri e della discussione che si fa nella Commissione di merito - in questo caso la Commissione bilancio - si esprime il parere finale per l'Assemblea. In questo caso, signora Presidente, non è stato possibile nemmeno dare il parere *ex post*, si sono sommate scorrettezze a scorrettezze. Per questa ragione, chiediamo alla Presidenza di valutare se non sia il caso di consentire alla Commissione affari europei di esprimere

Signor Presidente, sono lieto di poter dare la mia versione dei fatti, che risulta agli atti della riunione che abbiamo effettuato questa mattina sulla base di una decisione consensuale dell'ordine dei lavori della Commissione che era stato approvato, ai sensi del Regolamento e nei termini prescritti dal Regolamento, già nella giornata di ieri con programmazione del voto nella mattina di oggi con la convocazione di oggi mettendo al primo punto la discussione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. L'ordine dei lavori che abbiamo seguito è stato scrupolosamente attento al Regolamento, come ritengo di aver potuto sempre contribuire a fare, con l'aiuto dell'Ufficio di Presidenza e anche con l'atteggiamento di tutti i membri della Commissione, dove

Quando è stato avviato l'esame della NADEF questa mattina, diversi membri della Commissione hanno rilevato come l'esame di merito fosse già concluso

un valore unicamente formale, superfluo e vorrei dire praticamente inutile. Questo è il senso degli interventi che sono stati pronunciati

In questo senso, con l'atteggiamento che ho dovuto riscontrare che era quello di tutti, non si è proceduti al voto, com'era intenzione fare nella convocazione dei lavori della Commissione questa mattina. Quindi, non mi sento di poter confermare e riferire una testimonianza che sia corrispondente a quella che il senatore che ha preso la parola prima di me ha riferito. Questo per quanto riguarda la mia consapevolezza di ciò che è avvenuto in Commissione. Naturalmente, se ci fosse stata una richiesta di procedere al voto, questo era quanto era stato calendarizzato; quindi è stato per consenso che si è deciso di fermare lì la nostra attività, perché ormai superata, a giudizio di tutti, dall'esame della Commissione di merito, e di acquisire agli atti del verbale comunque lo strutturato parere presentato dal Capogruppo in Commissione del Partito Democratico. *(Applausi)*.

però a noi stamattina - lo segnalo - è stato detto che, poiché era stato già votato il parere dalla Commissione che aveva il compito di affrontare il tema, quindi dalla Commissione bilancio, sostanzialmente la la discussione sarebbe stata irrisoria e inutile nel poter modificare qualsiasi cosa. C'è stato anche un confronto, molto pacifico e tranquillo, tra me e il collega Borghi

hanno valore o no i pareri espressi dalle Commissioni? Perché se noi riteniamo che i pareri espressi dalle Commissioni hanno un valore per la Commissione competente a cui viene chiesto di lavorare su un testo, allora questi pareri devono essere depositati e discussi prima *(Applausi)*, altrimenti chiudiamo chiudiamo la saracinesca e diciamo alle altre Commissioni che non è importante che esprimano il parere, perché comunque può essere semplicemente un atto di testimonianza. Siccome noi facciamo i legislatori e non semplicemente coloro che portano testimonianza, direi allora che forse i due Presidenti della Commissione - che stimo e che fanno parte oltretutto della stessa forza politica - dovevano magari riuscire a confrontarsi sui tempi. Segnalo la Commissione politiche dell'Unione europea - lo dico con grande trasparenza e senza polemiche - ha stabilito di votare sempre nella mattinata di mercoledì, con con l'opposizione favorevole a questo, nostro malgrado, per venire incontro ai Commissari della maggioranza che sono impegnati in tante altre Commissioni, poiché in quella Commissione ci sono membri che spesso sono sostituiti. Quindi, si rischia che la maggioranza non abbia mai i numeri.

a non poter svolgere i lavori sempre a causa della maggioranza (davvero non lo voglio dire con spirito polemico, ma perché noi vogliamo fare il nostro lavoro), allora c'è un'ulteriore problema. Chiediamo quindi che i Presidenti delle Commissioni si parlino, che ai parlamentari venga consentito di svolgere il loro lavoro e che i senatori delle Commissioni competenti possano essere messi nella condizione di fare i senatori, che siano di maggioranza o di opposizione. Questo, cari colleghi, lo dobbiamo dire a garanzia di tutti, a garanzia del Paese che noi rappresentiamo.

per chiedere che la Presidenza venga formalmente investita della vicenda che oggi emerge nel corso di questa discussione, perché, a mio avviso, stanno cominciando a venire a galla due elementi strutturali che rischiano di inficiare la qualità della produzione legislativa di questo Parlamento. Un primo elemento è di carattere strutturale, cioè noi non ci stiamo rendendo conto che, in maniera subliminale, il combinato disposto fra la diminuzione del numero dei parlamentari (su cui preferisco non esprimere alcun giudizio) e la costante proliferazione del numero delle Commissioni, che mantengono il numero dei componenti previsto dal Regolamento precedente, sta creando oggettive condizioni di difficoltà ai lavori. Dico questo anche come elemento di solidarietà nei confronti dei colleghi della maggioranza, perché in questi casi l'opposizione ha la possibilità di astenersi o di svolgere una funzione quasi a corredo, mentre la maggioranza deve garantire il numero legale. Ritengo pertanto che ci sia un primo elemento da dover considerare, perché altrimenti andando avanti di questo passo non solo la qualità dei nostri lavori, ma anche la capacità di poter intervenire dal punto di vista della produzione legislativa rischia di essere denegata. A ciò si aggiunge il secondo elemento, signora Presidente, che io ravviso nelle parole molto forbite, ma politicamente estremamente preoccupanti del Presidente della 4a Commissione, che ha sostanzialmente tratteggiato l'idea che una Commissione parlamentare sia una sorta di orpello, una cosa sulla quale si può esprimere o non si può esprimere, si può votare o non si può votare, come se il voto, che è l'elemento discriminante, qualificante ed essenziale della nostra presenza di legislatori,

struttura legislativa di un Parlamento che è sempre più chiamato a ratificare, con buona pace della centralità parlamentare, e che non ha più una sua capacità propulsiva. *(Applausi)*. Questi due elementi incrociati producono la situazione che oggi è stata ravvisata, peraltro su un tema non del tutto banale come la NADEF, in cui evidentemente anche le indicazioni che ci stanno arrivando dal Fondo monetario internazionale indurrebbero una riflessione particolare, ma non voglio entrare nel merito della discussione che ci sarà successivamente (per noi interverrà il senatore Calenda). Tuttavia questi elementi inducono una riflessione dal punto di vista dell'impostazione dei nostri lavori, per cui le chiedo, signora Presidente, di investire la Presidenza di questi aspetti.

del voto sui pareri, dando per scontato che ormai non c'è più tempo. Questa è una violazione della prassi, forse minimale, ma che si va a inserire in un contesto in cui le prerogative del Parlamento vengono sempre più mortificate.

tutti ed è stata confermata da un *referendum* popolare che ha avuto quasi l'80 per cento di voti a favore e che non giustifica il fatto che poi non si adegui il Parlamento ed il suo Regolamento (alla Camera non è stato adeguato il Regolamento, al Senato qualcosa è stato fatto) e che quindi venga boicottata boicottata dall'interno in diverse maniere per dimostrare che è stato un errore. Questo è un tipo di propaganda che noi stigmatizziamo e vogliamo denunciare, perché non è la riduzione del numero dei parlamentari che sta affaticando i lavori del Parlamento, bensì una deriva che mina alla base la nostra democrazia e la rappresentanza popolare contro cui invece tutti dovremmo veramente combattere. Signor Presidente, credo che gli appelli al rispetto del ruolo del Senato siano sempre da ascoltare con attenzione, perché il nostro ruolo va preservato, sia che siamo in maggioranza, sia che siamo all'opposizione.

fare una cosa quando la Commissione ha deciso, senza opposizione al suo interno, *nemine contradicente*, di non dare il parere. Si può può esprimere, su questa decisione, un parere negativo o favorevole, ma di fatto non si può obbligare una Commissione ad andare contro la propria decisione, altrimenti veramente viene sminuito il ruolo della stessa. Certo, sarebbe più bello avere tanto tempo, ma alla luce della riduzione del numero dei parlamentari e della riduzione del numero delle Commissioni, la strada percorribile per avere dei lavori ordinati è precisamente quella che è stata scelta nella Commissione presieduta dal senatore Terzi di di organizzare i lavori in un certo modo, affinché ci si sappia regolare su quando si vota e su quando ci sono le discussioni, come si fa praticamente in ogni altro Parlamento. Noi abbiamo questa abitudine all'emergenza, per cui i nostri calendari dei lavori hanno una prospettiva di pochi giorni, ma un'organizzazione dei lavori è sicuramente una strada giusta.

che sicuramente va approfondita e se ne parlerà con il presidente La Russa, certamente sensibile a queste tematiche, ma non possiamo denunciare una prassi che è stata assolutamente corretta, seguita senza l'opposizione di alcuno, come se questa fosse una lesione del ruolo parlamentare.

scrupolosamente il Regolamento, però questo deve valere sempre e comunque. Quindi il nostro impegno è questo. Chiaramente per oggi è andata così, perché abbiamo anche tempi stretti e quindi il Presidente ha potuto fare

fare tra di noi perché ogni tanto anche un po' di autocritica penso non faccia male, altrimenti noi che siamo in maggioranza siamo sempre nel giusto e gli altri sbagliano sempre e viceversa. Ragionando così non riusciremo mai a trovare il giusto equilibrio che ci vuole in questi casi. Però, dall'altra parte, ricordiamo all'opposizione che lo stesso atteggiamento dovrà esserci quando le parti un domani - mi auguro il più lontano possibile - potranno essere invertite, perché tante volte questi discorsi si fanno sempre solo

ci si organizza, ci si mette d'accordo, si fa il possibile per seguire tutto, però evitiamo poi queste polemiche che in tanti casi rischiano di risultare anche un po' pretestuose. *(Applausi)*.

Presidenza, tenuto conto di tutti gli interventi. È ovvio che dal punto di vista strettamente formale e regolamentare, l'assenza di un parere ovviamente non inficia l'andamento dei nostri lavori.

dei rappresentanti della maggioranza. È evidente che è anche un problema di atteggiamento nell'organizzazione dei lavori. Essendo questa la determinazione di questa Presidenza, possiamo proseguire

a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla NADEF 2023. Questa Nota di aggiornamento rappresenta uno degli strumenti fondamentali sul ciclo di programmazione economica e finanziaria del Paese. L'articolo 7, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica ne prevede la presentazione alle Camere per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10-*bis* ne disciplina i contenuti. Per quanto riguarda innanzitutto il quadro macroeconomico tendenziale di riferimento, nel nuovo scenario la previsione di crescita del PIL per il 2023 viene corretta in via prudenziale al ribasso, passando allo 0,8 per cento rispetto all'uno per cento riportato nel quadro programmatico del DEF approvato nella scorsa primavera. Tale revisione dipende essenzialmente dall'imprevisto andamento negativo degli ultimi dati congiunturali, peggiore del previsto nella media del primo semestre rispetto a quanto stimato nel DEF 2023, e dall'incertezza sull'evoluzione del contesto internazionale anche rispetto agli ultimi fatti. Per il 2024, anche per via dell'effetto di trascinamento del rallentamento in corso, la revisione è più marcata, con la previsione di crescita del PIL ridotta all'uno per cento rispetto all'1,5 per cento, previsto sempre nel DEF, principalmente per il deterioramento del quadro internazionale. Nel biennio successivo invece la previsione di crescita resta invariata per l'anno 2025, confermando quanto ipotizzato ad aprile nel DEF ed è rivista marginalmente al rialzo per il 2026 (più 0,1 Questa nuova previsione macroeconomica tendenziale per il 2023 ed il 2024 è stata validata dall'Ufficio parlamentare di bilancio il 21 settembre scorso. Il quadro macroeconomico programmatico per gli anni 2024 e successivi, presentato in questa Nota, include l'impatto sull'economia delle misure che saranno adottate con la prossima legge di bilancio del 2024.

Le misure della manovra determinerebbero quindi rispetto allo scenario tendenziale un incremento del tasso di crescita del PIL di 0,2 punti percentuali nel 2024 e di 0,1 punti percentuali nel 2025. Il livello più alto del PIL, raggiunto nel 2025, unitamente all'esaurirsi degli effetti espansivi della manovra delineata, porterebbe ad una dinamica dell'attività meno accentuata nel 2026. Il quadro macroeconomico tendenziale per il 2023 e il 2024 è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nell'audizione del 9 ottobre scorso. Nella NADEF sono quindi presentate le previsioni di finanza pubblica basate sulla legislazione vigente aggiornate per il periodo 2023-2026. Esse indicano un percorso di costante miglioramento dell'indebitamento netto in rapporto al PIL per ciascuno degli esercizi considerati rispetto al precedente, ma, allo stesso tempo, un peggioramento delle previsioni rispetto a quelle del DEF 2023. Infatti, secondo questa Nota di aggiornamento, le previsioni a legislazione vigente vedranno un miglioramento del rapporto indebitamento netto-PIL, che, partendo dall'8 per cento del consuntivo 2022,

L'andamento tendenziale stimato da questa Nota riflette un costante miglioramento del saldo primario, tale da compensare il peggioramento della spesa per interessi. Inoltre, la revisione delle previsioni della NADEF rispetto a quelle del DEF sconta la riclassificazione delle spese per il superbonus per interventi sostenuti negli esercizi 2024 e 2025. Infine, si nota che, come evidenzia specificatamente la NADEF, all'interno del quadro di finanza pubblica è confermata la piena attuazione dei programmi di spesa finanziati dal dispositivo per la ripresa e resilienza.

Gli spazi finanziari che si rendono disponibili quale differenza tra gli andamenti tendenziali e programmatici aggiornati, che includono anche la maggiore spesa per interessi passivi conseguenti al maggior disavanzo, sono pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi del 2024 e a 4,6 miliardi nel 2025. Nel 2026, invece, il saldo obiettivo implica una correzione di 3,8 miliardi di euro rispetto all'indebitamento netto tendenziale, che consente di riportare lo stesso al di sotto della soglia del 3 per cento. Secondo quanto esposto nella Nota, la manovra di finanza pubblica per il 2024-2026 continuerà ad essere orientata a principi di prudenza, cercando di contemperare l'obiettivo di fornire sostegno all'economia attraverso misure mirate con l'obiettivo di assicurare il rientro del *deficit* al di sotto del 3 per ed un percorso di riduzione credibile e duraturo del rapporto debito-PIL. In coerenza con le raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea per l'Italia, si intende ritirare gradualmente le misure di sostegno connesse agli aumenti dei prezzi dei beni energetici. Con la prossima manovra di bilancio, il Governo continuerà a sostenere la domanda privata e a contrastare il calo del potere di acquisto delle retribuzioni causato dall'inflazione, attraverso interessi mirati. La dinamica degli interessi passivi prospettati in questa Nota mostra un significativo incremento del peso degli interessi sul PIL, che passerebbero dal 3,8 per cento del PIL del presente anno al 4,2 nel 2024, per raggiungere il livello per cento nel 2026. In rapporto alle stime recate dal DEF 2023, l'aumento è comunque contenuto per ogni anno in 0,1 punti percentuali di PIL, in virtù dell'elevata durata media del debito pubblico, che consente di smussare nel tempo l'impatto del rialzo del tasso di interesse. Il saldo primario mostra un deciso miglioramento per il 2023, attestandosi all'1,5 per cento del PIL, rispetto al 2022, quando il medesimo aggregato si collocava al 3,8 Nel 2024 si prevede un ulteriore miglioramento, che porterebbe il saldo primario a -0,2 per cento. Esso diverrebbe poi positivo a partire dal 2025, per raggiungere l'1,6 per cento nel 2026. Ad un confronto con il DEF della primavera scorsa, i saldi primari per il periodo in esame risultano comunque in riduzione di circa 0,5 punti percentuali per ogni anno considerato. Con riferimento all'indebitamento netto strutturale, il quadro programmatico delinea un percorso di riduzione più morbido rispetto a quello previsto nell'ultimo DEF. Il processo di riduzione del debito pubblico, poi, si dovrebbe collocare lungo una traiettoria leggermente più ripida. Stante la sostanziale stabilità del rapporto debito-PIL, intorno al 140 per cento in tutti gli anni di riferimento, il quadro programmatico ora definito lo vede leggermente ridursi per cento del 2023 al 139,6 per cento del 2026, a fronte della sostanziale stabilità scontata nel quadro e di un calo più pronunciato, ma partendo da valori più elevati, sulla base del quadro programmatico del DEF di aprile. La NADEF segnala peraltro che la dinamica soltanto lievemente decrescente del rapporto debito-PIL nello scenario programmatico sopra delineato tiene conto di una serie di fattori che verosimilmente eserciteranno una spinta al rialzo del rapporto: le prolungate incertezze nel contesto geopolitico, che influiranno negativamente sulla crescita economica; il tasso di inflazione in discesa, che attenuerà la spinta al PIL nominale; il recepimento dei maggiori tassi di rendimento da parte di una quota crescente dei titoli debito, che spingerà al rialzo la spesa per interessi complessiva; il flusso dei crediti di imposta relativa agli incentivi per *bonus* edilizi utilizzati in compensazione, che rilevano ai fini della contabilizzazione del debito pubblico in base al profilo di cassa della loro effettiva fruizione. Alla Nota di aggiornamento risultano allegati: la nota illustrativa sulle leggi pluriennali di spesa in conto capitale a carattere non permanente; il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali; il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva; la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva. Unitamente alla NADEF, il Governo ha trasmesso al Parlamento la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio Grazie scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT). In ordine alla sussistenza dei previsti presupposti per intervenire, si sottolineano i segnali di frenata nella crescita del PIL registrati a partire dai mesi primaverili dell'anno in corso, che non devono essere trascurati, anche se determinati da fattori esogeni rispetto all'economia nazionale. Inoltre, si teme che lo scenario macro finanziario possa ulteriormente deteriorarsi a causa dell'eccessivo prolungarsi della fase di inflazione, che indurrebbe le principali banche centrali ad inasprire le politiche monetarie, o di un ulteriore rallentamento delle principali aree economiche che solitamente trainano il commercio mondiale. Incombe anche il rischio, a livello geopolitico, di un acuirsi delle attuali tensioni internazionali, che potrebbero dare luogo a nuovi *shock* ai prezzi dell'energia oppure a restrizioni nella catena di offerta in settori strategici per l'economia. Il Governo presenta quindi la richiesta di un margine di manovra in termini di indebitamento da utilizzare per adottare provvedimenti che si ritengono in grado di fornire un sostegno all'economia nel breve termine, quali la riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori e un primo intervento attuativo della delega fiscale, al fine di trasformare, in prospettiva, il sistema tributario in un fattore di crescita e di sviluppo. Con la Relazione in oggetto, sentita la Commissione europea, il Governo chiede l'autorizzazione alla revisione degli obiettivi programmatici di indebitamento netto previsti nel DEF 2023 per un importo, in termini percentuali di PIL, pari allo 0,8 per cento nel 2023, allo 0,6 per cento nel 2024 e allo 0,4 per cento nel 2026. Le risorse relative al 2023 saranno destinate, attraverso un provvedimento d'urgenza delle prossime settimane, al conguaglio anticipato dell'adeguamento Istat per i trattamenti pensionistici previsti per l'anno 2024, a misure per il personale delle pubbliche amministrazioni e alla gestione dei flussi migratori. Nel 2024 e nel 2025 le risorse saranno utilizzate nell'ambito del prossimo disegno di legge di bilancio per il taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024; all'attuazione della prima fase della riforma fiscale; al sostegno alle famiglie e alla genitorialità; alla prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità; al potenziamento degli investimenti pubblici, con priorità per quelli previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché al finanziamento delle politiche invariate. Il livello del saldo netto da finanziare del bilancio dello stato di competenza potrà aumentare fino a 202,5 miliardi nel 2024, a 168 miliardi nel 2025 e a 134 miliardi nel 2026.

Le tre raccomandazioni del Consiglio vertono rispettivamente su tre aspetti: perseguimento di una politica di bilancio prudente e di supporto alla crescita sostenibile; accelerazione dell'attuazione del PNRR, di REPowerEU e dei programmi della politica di coesione; promozione della sostenibilità ambientale. All'interno della Parte IV della NADEF il Governo illustra le iniziative politiche normative e amministrative finora intraprese al fine di adempiere alle suddette raccomandazioni. conclusione, Presidente, la NADEF 2023 reca l'elenco dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica 2024-2026, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorre al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In particolare, sono dichiarati collegati alla manovra di bilancio 32 disegni di legge, cinque dei quali già presentati e in corso d'esame presso

Informo l'Assemblea che l'esame del documento si concluderà con l'approvazione di due distinti atti di indirizzo: il primo, relativo alla relazione di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, 243 del 2012, da votare a maggioranza assoluta; il secondo, relativo alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, da votare a maggioranza semplice. Le proposte di risoluzione ad entrambi i documenti dovranno essere presentate entro la fine della discussione. Dichiaro aperta

in una struttura di *deficit* ordinaria dopo anni di *deficit* straordinari, perché legati a eventi straordinari, dal Covid alla guerra. in questo condivido in pieno la diagnosi del Governo - che dovete confrontarvi con quello che, a nostro avviso, è stato il più grande disastro delle finanze pubbliche della storia repubblicana recente, che si chiama superbonus. Voglio premettere tutto questo per dire che non partiamo, come non siamo partiti l'anno scorso, con un'idea preconcetta. Anzi, ricorderete che l'anno scorso sulla legge di bilancio abbiamo riconosciuto la responsabilità del Governo e abbiamo avviato un confronto. Allo stesso modo, però, oggi dobbiamo dire che questa NADEF disegna un quadro di finanza pubblica, prima di tutto, irrealistico e, in secondo luogo, molto pericoloso, perché adottato nel mezzo di una doppia crisi geopolitica, con una situazione che rimane straordinaria. Parto da un dato: non ci sarà l'1,2 per cento di crescita. Questa è una presa in giro che ci possiamo raccontare in quest'Aula e che è buona per un paio di *talk show* televisivi. Il consenso

Da parte nostra, dunque, il punto non è la difficoltà della situazione che vi trovate ad affrontare, ma il modo in cui la state affrontando. Noi nel 2026 arriveremo a 104 miliardi di euro di servizio al debito: è un numero gigantesco e impressionante, che forse tutti stiamo sottovalutando. Come si fa in queste condizioni a prevedere, su 15,7 miliardi di *deficit* extra, 14 miliardi di tagli di tasse temporanei, operati di

delle famigerate clausole IVA, facendo indebitamento in *deficit*, in alcuni casi - penso alla delega fiscale - con un impatto assolutamente ininfluente sui salari bassi, da 8 a 20 euro.

In aggiunta a questo, ci sono 2 miliardi di tasse sugli extraprofitti. Stendo un pietoso velo su quello che è avvenuto a proposito della tassa sugli extraprofitti bancari, che è stata prima annunciata, poi modificata in serata e infine modificata nuovamente, con un gettito al momento decisamente sovrastimato. Noi riteniamo inoltre che ci sia un problema di costituzionalità: gli scostamenti di bilancio si fanno per le emergenze. Che emergenza è tagliare provvisoriamente le tasse? È una questione strutturale, non emergenziale. Dunque c'è una questione che ha a che fare con un problema di costituzionalità di quello che vi apprestate a chiedere al Parlamento. Cosa si poteva fare? Noi siamo abituati a dire cosa si poteva fare. Si poteva fare una cosa di buon senso: iniziare a rimettere in piedi i pilastri scossi dei nostri diritti sociali. Siamo diciassettesimi per investimenti sulla sanità in Europa e venticinquesimi sulla scuola.

Non ci sono i 10 miliardi? Okay, ma ne mettiamo almeno quattro, cioè quelli che le Regioni chiedono, altrimenti va tutto a pezzi? I numeri sono talmente impietosi che li possiamo ricordare qui: 10 milioni di prestazioni urgenti arretrate, 4 milioni di persone che non si curano. Invece facciamo finta di niente e diamo 20 euro in più al mese a una persona che magari ha un genitore anziano che va curato a spese proprie. Ma che senso ha, che logica ha tutto questo? C'è l'annosa questione di non aver preso le risorse del MES sanitario, uno dei grandi delitti che questo e altri Governi hanno compiuto. *(Applausi)*. Perché non si negoziano la ratifica del MES e la riapertura di una linea di MES sanitario per poter attingere a costi più bassi?

non mi spiego perché non riusciamo a fare cose che sono semplicemente di buon senso. C'è un problema sui salari? Certo che c'è, ma allora perché non si può fare il salario minimo, come abbiamo proposto, a 9 euro? a 9 euro? Ho l'impressione che, alla fine della fiera, quello che sta succedendo è che ci prepariamo a vedere una manovra e una legge di bilancio fondate su qualche mancia provvisoria, mentre tutto il resto si sgretola. Rivendicherete queste mance provvisorie, siete i primi a farlo, tuttavia alla fine ci sarà la continuazione di un declino italiano che è fatto di questo: pilastri della Repubblica che si sgretolano (sanità, scuola); modello di sviluppo fondato su salari bassi; tagli di tasse provvisori che poi rientrano per cui la pressione fiscale complessiva non varia. Questa è la storia della Seconda Repubblica. Voi siete su quella traccia non sarebbe così grave - perché è la storia della seconda Repubblica - se non fosse che siamo davanti a un periodo in cui il mondo è in fiamme;

Cari colleghi, oggi affrontiamo uno dei documenti più importanti, che delinea sicuramente la rotta che questo Governo vuole intraprendere. Purtroppo, a noi sembra che questa rotta ci porterà presto a sbattere. Lo scorso anno vi avevamo avvisato, vi avevamo detto che stavamo andando in una direzione sbagliata sbagliata e che le misure politiche prese avrebbero portato questi risultati. Siamo stati facili profeti, non volevamo esserlo, però era prevedibile: se bloccate le imprese, bloccate i crediti, tagliate i consumi, c'è un'inflazione alle stelle promettete il taglio delle accise e non lo fate, capite che tutto quello che avete fatto è il risultato del deterioramento dei dati macroeconomici di questo Paese. Infatti, se vedete, c'è una decrescita della produzione, abbiamo un carovita pazzesco e non si riesce più a comprare nulla (anche questo bollino che avete messo io non l'ho visto da nessuna parte, ma non sta dando i risultati sperati). Tutto quello che avevamo detto lo scorso anno

quindi che ci siamo messi in un quadro macroeconomico assolutamente pericoloso e purtroppo, anche le previsioni che fate per il 2025 e il 2026 sicuramente verranno riviste al ribasso. Qual era la strada che noi avevamo dettato - e potete verificarlo - lo scorso anno? Anch'io in questa sede parlai proprio di questo documento. Sicuramente non erano i 1.000 euro con un *click*; noi avevamo detto dove trovare i soldi e dove spenderli. Dove trovare i soldi? Sicuramente negli extraprofitti. Ci avete riempito le orecchie per mesi dei fannulloni, allora ditemi voi: chi sono i fannulloni? mantiene un tasso di interesse basso sui conti correnti e aumenta in maniera vertiginosa quello che dà a prestito e realizza un extraprofitto senza fare nulla, stando comodamente seduto sul divano? divano? Tutte quelle banche che hanno fatto questo hanno guadagnato miliardi di euro *(Applausi)*, non le poche centinaia di euro del povero cristo. Perché quelli là non dite che sono dei fannulloni, delle persone che sul divano hanno fatto miliardi di euro?

Quando le aziende petrolifere hanno fatto miliardi di euro senza fare nulla, perché avevano contratti pluriennali a un prezzo basso stabilito e poi hanno guadagnato miliardi di euro stando comodamente sul divano, quelli non sono fannulloni? Allora, signori miei, queste aziende hanno giustamente diritto a un profitto, ma non a fare miliardi senza fare nulla, senza un po' di lavoro. Mi dispiace che sia andato via il senatore Calenda, perché almeno le imprese del superbonus hanno restaurato mezzo milione di case. Se li sono guadagnati i soldi perché hanno faticato e fare un immobile è sudore, non come quelli degli extraprofitti che hanno fatto miliardi di euro non facendo nulla. Lì dovevate tassare: c'erano almeno 10 miliardi da prendere sugli extraprofitti e non l'avete fatto, perché sono amici. sono amici. Lì c'erano i soldi da prendere e quei dieci miliardi dove li potevamo spendere, cari colleghi? Semplicemente abbassando le accise, come avevate promesso, magari sul trasporto di merci, perché se avessimo abbassato le accise sul trasporto delle merci, probabilmente il carrello della spesa non sarebbe arrivato a questi livelli. Vi avevamo detto quindi sia dove prendere i soldi, sia dove utilizzarli, ma non l'avete fatto ed è ridicolo quello che avete fatto con le banche. Avete promesso appunto gli extraprofitti e poi è sparito tutto. Scusate, voi dove volete fate cassa, sul povero cristo che prende 400 euro al mese di reddito di cittadinanza, che sono appena 10 o 15 euro al giorno, su chi ha fatto miliardi di euro speculando sull'aumento dei tassi di interesse e sull'aumento dei prezzi energetici? Ditemi voi cos'è più equo. Dove volete prendere quei soldi: da chi ha fatto miliardi di speculazione sull'aumento dei tassi di interesse o sul povero cristo che non arriva a fine mese? Di questo vi dovete rendere conto, perché c'era dove prendere i soldi. C'erano i soldi per sistemare i tanti problemi che abbiamo

ma c'è chi ha fatto miliardi su questi aumenti dei prezzi, sull'aumento dei tassi d'interesse e sull'aumento dei prezzi energetici; c'è chi ha fatto miliardi di extraprofitti e a loro dovevamo dire, se sono veramente aziende patriote: patriote: hai fatto miliardi su quegli extraprofitti? Dammene una parte, perché devo sistemare i problemi che ci sono in questo Paese. Penso, ad esempio, ai mutui, che le persone non riescono più a pagare, o anche

un errore gravissimo non concedendo la proroga, perché ormai il *budget* del superbonus è quello e non può aumentare. Se voi non concedete la proroga, fate sì che le aziende debbano accelerare il lavoro e finire tutto nel 2023 e in questo caso le aziende scaricheranno il costo nel 2024. La proroga conviene al bilancio dello Stato, perché le aziende prendono tempo, realizzano i lavori nel 2024 e in questo modo scaricano il costo nel 2025.

PIL; il rapporto tra deficit e PIL è migliorato col superbonus. State andando invece in una direzione completamente sbagliata, state distruggendo l'economia e indebitando il Paese. Almeno una delle due: o fate crescere l'economia e indebitate il Paese, oppure riduciamo il debito e distruggiamo l'economia. Voi invece state facendo un doppio danno, state prendendo il peggio del peggio e state andando in una direzione che ci porterà a sbattere.

che portano i soldi nei paradisi fiscali. Non colpisce i ricchi, quelli che hanno guadagnato dall'aumento dei tassi di interesse, ma i poveri.

con questi errori non sbattete solo voi come maggioranza, perché già le imprese che vi hanno votato non vi vogliono più vedere, soprattutto quelle del settore edile; sbatterà tutto il Paese, sbatteremo anche noi, i nostri figli e le nuove generazioni che sono qui, che chiedono un futuro soprattutto per l'emergenza climatica in atto. Sbattiamo tutti, quindi i danni che state facendo con questa NADEF poi li paghiamo tutti.

questa sede per il suo reale pragmatismo, che ci fa comprendere perfettamente la situazione economica e finanziaria, ma anche quella geopolitica in cui ci troviamo. La crisi mediorientale, con la brutale aggressione di Hamas contro Israele, aggiunge instabilità a un quadro già particolarmente complicato, fatto di conflitti di intensità variabile, tensioni mai sopite e un mutato scenario geopolitico, del quale ancora non si riesce a tracciare un contorno ben definito. Il conflitto in Ucraina, la già citata crisi del Medio Oriente, il conflitto in Nagorno-Karabakh, le tensioni dell'Indopacifico - sulle quali mi permetta, signor Presidente, di fare una piccola riflessione: occorrerebbe probabilmente prestare a queste situazioni una maggiore attenzione - l'instabilità poi del Nord Africa e del Sahel dietro a tutte queste situazioni, azioni di interferenza di potenze ostili volte a destabilizzare non solo il nostro Paese, ma anche l'Europa e l'Occidente intero, ci fanno evidentemente capire che stiamo vivendo un momento delicato che aggiunge incertezza e instabilità.

puntando anche a un contenimento dei costi dell'inflazione e alla sostenibilità dei conti pubblici, rafforzando la fiducia degli investitori. aspetti invece meno positivi - non evidentemente da imputare a questo Governo, ma ad altri attori - sento il dovere di constatare come le scelte politiche restrittive prese a livello europeo per contrastare l'inflazione abbiano sottratto alla disponibilità del Governo importanti risorse che avrebbero invece potuto essere investite e destinate a specifiche politiche e operazioni di sviluppo. Per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica, l'aumento dell'indebitamento netto, ascrivibile a scelte scellerate del passato, come il superbonus, che ancora qualcuno, anche in quest'Aula, vuole difendere. Come ricordato dal ministro Giorgetti, in assenza di questa contabilizzazione, l'Italia avrebbe certamente raggiunto l'obiettivo prefissato e qui farò saltare qualcuno sulla sedia riportando un dato significativo. Oggi i nostri imprenditori, nell'epoca della transizione ecologica, pagano le quote di emissione di CO2 circa 90 euro a tonnellata. Ebbene, pensate che l'operazione invece, è costata allo Stato oltre 500 euro a tonnellata. La misura è quindi anche poco *green* rispetto ad altri investimenti possibili e capisco qui perfettamente, visto che è stato riportato poc'anzi, l'allora ministro Cingolani, che secondo me i conti li sa fare molto bene, che era assolutamente contrario a prolungare il superbonus, proponendo invece una detrazione - altrettanto appetibile, Permettetemi infine, da cittadino del Friuli-Venezia Giulia, Regione a Statuto speciale, dove l'autonomia differenziata è una realtà, di auspicare che nel più breve tempo possibile questa importante riforma dia compimento a quanto già previsto dal Titolo V della Costituzione. Anche questo epocale passaggio permetterà allo Stato una migliore gestione programmatoria e ai territori di essere finalmente decisori,

come lo è stato il ministro Giorgetti, come lo siamo noi della Lega e come lo è questo Governo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, la Nota di aggiornamento 2023 sulle previsioni economiche e finanziarie che ci è stata sottoposta ruota intorno a due concetti importantissimi: prudenza e responsabilità. Le previsioni della NADEF sono compatibili con gli andamenti macroeconomici, hanno un riscontro con i dati reali e soprattutto tengono conto della situazione dei conti e dei provvedimenti che abbiamo ereditato, come il conto che ci è stato lasciato da pagare con il superbonus. Il documento oggetto di discussione quest'oggi rappresenta un atto di rispetto verso i nostri cittadini e le generazioni future. Le parole d'ordine, come detto, sono prudenza e responsabilità. Ma quando parlo di prudenza e soprattutto di responsabilità a cosa mi riferisco? Innanzitutto, basta con provvedimenti e misure che sperperano soldi senza raziocinio, causando buchi, per non dire voragini, nei conti pubblici. Il nostro operato invece deve essere guidato verso un disegno ampio, che guarda un orizzonte non nel breve termine, come se fossimo in campagna elettorale, ma nel lungo termine, che mira a manovre ambiziose che impongono oculatezza, buon senso e razionalizzazione delle risorse. Parlando di buon senso e scelte per il benessere della collettività, la NADEF conferma *in primis* il taglio del cuneo fiscale e l'applicazione della delega fiscale per proseguire nella politica di riduzione delle tasse, così come restano l'aiuto ai redditi medio bassi, la decontribuzione già decisa l'anno scorso e gli interventi a favore delle famiglie con figli. Inoltre, prosegue il lavoro sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego, in particolare nel comparto della sanità. Certo, in generale, se lo analizziamo, il quadro mondiale si presenta molto vario e anche con una prospettiva economica globale condizionata da alcuni fattori quali la persistente elevata inflazione, le condizioni finanziarie più restrittive, le tensioni geopolitiche, le restrizioni agli scambi internazionali, l'insicurezza energetica e quella alimentare, i livelli più elevati di debito e i correlati rischi per la stabilità finanziaria. L'economia italiana ovviamente, come l'intera eurozona, ha risentito dell'indebolimento del quadro globale, che ha leggermente rallentato la crescita e la spinta dei primi mesi dell'anno. Ci sono alcune note positive che si possono interpretare per le previsioni per il 2024. Infatti, nonostante l'elevata inflazione e il rallentamento del ciclo economico in corso, nella prima parte del 2023 si sono registrati una diminuzione del numero di soggetti disoccupati e un aumento degli occupati. Ad agosto l'occupazione torna a crescere, segnando +59.000 unità rispetto al mese precedente. Il tasso di occupazione sale al 61,5 per cento e ad agosto il tasso di disoccupazione totale scende al 7,3 per cento. Quali sono quindi le strategie che vogliamo utilizzare? Occorre innanzitutto razionalizzare le spese. Importantissima è poi la riforma fiscale, infatti rispetto ad essa il Governo ha riportato la descrizione dei contenuti della delega fiscale approvata dal Parlamento il 4 agosto scorso. Questa prevede quale obiettivo fondamentale la semplificazione del sistema tributario, la riduzione delle aliquote Irpef e dei relativi scaglioni, preservando il principio di progressività, al fine di ridurre il carico fiscale sul lavoro e promuovere l'equità orizzontale, nonché la progressiva rimodulazione o eliminazione di alcune agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi. Viene inoltre ribadito l'intendimento di ridurre nel 2024 il cuneo fiscale sui lavoratori. E ancora, abbiamo le misure del PNRR. Infatti, per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e basti far sapere all'opposizione e ai detrattori del Governo e della maggioranza che la terza rata che ammonta a circa 18,5 miliardi è stata appena erogata. Questo fa capire che, al di là dei dubbi pronostici dell'opposizione e di chi vuole male al Governo e ai cittadini, se si lavora con impegno e con incessante senso di responsabilità nei confronti della cittadinanza, i risultati si ottengono. Questo riconoscimento da parte dell'Europa è il prodotto di un duro lavoro, volto a raggiungere obiettivi complessi nei settori della concorrenza, della giustizia, dell'amministrazione pubblica e fiscale, dell'istruzione, del mercato del lavoro e del sistema sanitario. Questo pagamento non coprirà solo gli investimenti per sostenere la transizione digitale e verde, ma promuove anche la ricerca, l'innovazione e l'istruzione. È un passo significativo verso un futuro migliore e più sostenibile.

Le previsioni tendenziali della NADEF indicano un percorso di costante miglioramento dell'indebitamento netto in rapporto al PIL: si passa dal 5,2 per cento del 2023 Pertanto, è vero che ad oggi l'indebitamento è stato aumentato, ma - come detto in precedenza - è stato necessario a causa anche e soprattutto del superbonus, un provvedimento sul quale economisti e osservatori concordano sia stato eccessivamente generoso e abbia finito per gravare in modo eccessivo sulle casse dello Stato. Grazie al superbonus questa programmazione è nettamente sottotono rispetto a quella che sarebbe dovuta e potuta essere. Per citare il *premier* Giorgia Meloni è «il male che non consentirà a questa legge di bilancio di volare alto». Per quanto riguarda invece il comparto dell'agricoltura, visto il valore strategico che il settore agricolo riveste per la nostra economia, che solo l'anno scorso ha generato un valore aggiunto di 38,5 miliardi di euro, la Nota di aggiornamento conferma l'impegno del Governo nel forte sostegno al nostro settore primario. Si prosegue, è un duro lavoro già cominciato nella scorsa legge di bilancio. È stato infatti pubblicato in agosto il provvedimento che sblocca le risorse previste dalla legge di bilancio 2023 per sostenere l'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura; 75 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Si dà così continuità a quanto già programmato. L'importanza della programmazione è cruciale per raccogliere le sfide e le opportunità che ci si presentano davanti e per stare al passo con i tempi. Le tecnologie digitali avanzate nell'ambito agricolo svolgono un ruolo essenziale nel supportare gli agricoltori nelle loro attività quotidiane e nella pianificazione delle strategie strategie aziendali. Grazie a queste soluzioni innovative e all'impiego delle tecnologie digitali, le aziende agricole possono migliorare la redditività e promuovere la sostenibilità economica, ambientale e sociale nelle loro operazioni. Inoltre, queste tecnologie favoriscono la creazione di un ciclo virtuoso che genera valore non solo per l'azienda agricola stessa, ma anche per tutti gli attori della catena di produzione agricola, creando così un impatto positivo su tutta la filiera. Vi garantisco che uno dei settori che trae notevoli benefici da questa innovazione è sicuramente l'agricoltura, spesso purtroppo considerata conservatrice poco incline al cambiamento, ma che negli ultimi anni sta sperimentando con successo il potenziale della digitalizzazione, con risultati tangibili e facilmente misurabili. Il nostro obiettivo è trasformare l'agricoltura italiana in un'agricoltura 4.0, con un minor uso di pesticidi. Importantissimo è stato l'emendamento sulle tecniche di evoluzione assistita, perché permette di sperimentare in campo delle piante più resistenti ai cambiamenti climatici e alle esigenze ambientali. In un panorama globale caratterizzato da complicati dilemmi economici e politici, con l'onere di una massiccia eredità di problemi amministrativi lasciati dalle gestioni precedenti, il Governo attuale persiste instancabilmente nel suo impegno di indirizzare risorse strategiche verso i cardini irrinunciabili che costituiscono il fondamento della nostra Nazione: famiglia, lavoratori e imprese; scelte coraggiose e ambiziose che non siano basate sullo sperpero di denaro pubblico, in barba ai conti e senza un minimo di responsabilità verso i nostri cittadini. Noi vogliamo fare scelte di buon senso che abbiano come obiettivo la ripresa economica del Paese e il rilancio della nostra economia. Vogliamo programmare e non mettere una pezza per le emergenze o promuovere provvedimenti di dubbia autorità per poi dover fare i conti con i buchi e le voragini di spesa. Noi vogliamo che l'Italia cresca, che prosperi, che intraprenda un cammino di crescita che possa dirsi strutturale e per tutto il sistema Italia. Questo è quello che sta facendo il Governo Meloni. Questo è quello che ci hanno chiesto i nostri elettori.

Rispetto appunto alle previsioni di aprile, che scontavano già le variabili esogene che pesano su tutta l'economia mondiale, si sono aggiunte ora ulteriori variabili. avuto l'aumento del costo dell'energia e delle materie prime, che ovviamente incide anche sul costo dei prodotti lavorati e quindi sulle nostre esportazioni; successivamente abbiamo avuto un aumento dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, prima la Federal Reserve in America e poi la Banca centrale europea. Ora si è profilato un nuovo conflitto tra palestinesi e israeliani, che non sappiamo ancora come coinvolgerà il Medio Oriente, ma che ha già avuto un ulteriore impatto negativo sui prezzi del petrolio e del gas. In questo quadro si decide di utilizzare maggiore indebitamento, facendone richiesta al Parlamento, un quadro veramente eccezionale, perché con l'aumento dell'inflazione le famiglie hanno perso potere di acquisto e le aziende hanno ridotto la loro propensione agli investimenti. Riduzione dei consumi e contrazione degli investimenti portano a evidenti effetti negativi sulla nostra economia. Le conseguenze che gli eventi bellici creano sui prezzi dell'energia, delle materie prime e dei prodotti al consumo sono certamente eccezionali; così come eccezionali sono un'inflazione arrivata fino all'11 per cento (ora in discesa, ma su livelli ancora troppo alti), e tassi di interesse, conseguenti al rialzo del tasso centrale della BCE, che penalizzano il credito alle famiglie e alle imprese. Ed è eccezionale il rallentamento del ciclo economico che ne consegue. Peraltro, queste risorse a debito vengono in larga parte utilizzate proprio per misure che sostengono il potere d'acquisto delle famiglie italiane. Ecco riassunto il motivo per cui il Gruppo Forza Italia voterà a favore della relazione che chiede lo scostamento di bilancio. Va sottolineato, inoltre, che si tratta di un momento di grande incertezza su tutte le economie mondiali. E questo dato viene segnalato anche dai rendimenti dei titoli di Stato (non solo quelli italiani), soprattutto quelli a due anni. I rendimenti dei buoni italiani e dei *treasury* americani hanno prima superato e ora sono a ridosso del 5 per cento. Il rendimento dei titoli a trent'anni, simile a quello italiano, è al momento inferiore a quello dei titoli a due anni, segno di un'incertezza generale nel breve periodo che condiziona tutti gli investitori. All'Italia, inoltre, conviene indebitarsi ora che il costo medio del debito è più basso della crescita nominale, usando l'indebitamento per aiutare la crescita economica. La soluzione è quindi far crescere la nostra economia, proprio perché uno *stock* di debito così elevato esige una crescita sostenibile. La spinta maggiore alla crescita del PIL deve venire - e ne siamo convinti verrà - dagli investimenti. Sappiamo che gli investimenti sono legati soprattutto al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ecco perché tutte le risorse europee, quelle del PNRR, quelle del REPowerEU e quelle dei fondi europei, vanno ottimizzate e spese meglio, affinché realizzino il più alto moltiplicatore. Allo stesso tempo, è necessario stabilizzare i saldi di finanza pubblica verso valori più sostenibili. Quindi il controllo ferreo sui conti pubblici e la revisione della spesa, eliminando gli sprechi, sono il modo più appropriato per mettere in fila i numeri nella prossima legge di bilancio. bilancio. Le due azioni volte a massimizzare il risultato delle risorse europee, attraverso gli investimenti e il percorso di sostenibilità dei conti pubblici, possono rafforzare la fiducia dei mercati e degli investitori. innanzitutto valorizziamo il ruolo degli investimenti pubblici, anche investendo nelle reti stradali e nelle reti ferroviarie. Un tema che si è toccato molto è la questione dei bonus. Ebbene, messi da parte i *bonus* troppo generosi e dai crediti incontrollabili, che hanno generato un punto di PIL di indebitamento netto nel solo 2023, dobbiamo però continuare a sostenere l'edilizia in altri modi, trovando nel contempo soluzioni ai ai problemi lasciati sul tappeto dal 110 per cento. Penso, ad esempio, alla doverosa proroga di qualche mese per consentire la fine dei lavori e la chiusura di questo 110 Allo stesso tempo, va rafforzata la coesione sociale. Pertanto, le misure che il Governo ha tratteggiato e ha annunciato che verranno inserite nella legge di bilancio 2024 mirano a trovare il sostegno, non solo dei cittadini, ma anche delle parti sociali. Poi si dovranno affrontare i problemi cronici della nostra economia, ma proprio il fatto che alla decisione di bilancio siano allegate trentuno riforme da approvare con altrettanti disegni di legge va nella giusta direzione. La risposta migliore è attuare quelle riforme, che seguono le raccomandazioni europee e servono a garantire chi guarda all'Italia per investire. Ecco perché condividiamo i contenuti e le indicazioni della NADEF, seppur ancora sommari rispetto a un quadro che si sta riempiendo in vista della legge di bilancio. La NADEF annuncia una manovra realista, concreta e allo stesso tempo prudente. Ci complimentiamo, quindi, con il ministro Giorgetti e con il Governo, per l'ottimo approccio che hanno dato alla decisione di bilancio per il prossimo triennio attraverso la Nota di aggiornamento al DEF. Presidente, io ho una visione di come sta andando l'economia del nostro Paese diametralmente opposta a quella di chi mi ha preceduto. Avevamo già detto durante la discussione dello dello scorso anno, soprattutto sulla legge di bilancio, che non c'erano visione e misure di rafforzamento del sistema economico del Paese e di promozione dell'impresa e che questo avrebbe portato a una contrazione della crescita. È facile essere Cassandre quando si sanno leggere i provvedimenti che arrivano da questo Governo. Come avevamo previsto, così è stato. Tant'è che questa Nota di aggiornamento si preannuncia

Come a dire: dagli errori del passato non abbiamo imparato niente e continuiamo a ripeterli continuamente, a spese dell'Italia e dei cittadini italiani. *(Applausi)*. Io mi occupo prevalentemente di sanità e, se guardiamo i dati della NADEF riguardo alla sanità, non possiamo che davvero metterci a piangere. Dopo che, finalmente, nella scorsa legislatura, con i Governi Conte, avevamo invertito la rotta di definanziamento della nostra sanità, che andava avanti da un decennio, se non di più, abbiamo ripreso di nuovo la stessa china pericolosa. Gli allarmi arrivano da più parti e restano puntualmente inascoltati. Finanziamento: per il 2024, 6,2 per cento del PIL; per il 2025, 6,2

che non faceva presagire niente di buono. Chi è arrivato ha sbraitato per anni in quest'Aula contro Draghi e sta facendo peggio di lui. Mi si dice che non bisogna guardare il rapporto rispetto al PIL. Allora guardiamo la spesa *pro capite* della nostra sanità. In Italia si attesta a circa 3.200 dollari *pro capite*. La media OCSE è pari a 3.899, la media europea a 4.128. Non aspiriamo certamente ai livelli della Germania, che supera i 6.000 dollari *pro capite*. Noi aspiriamo sempre al peggio e non andiamo sicuramente verso una direzione migliore. I problemi della nostra sanità li conosciamo tutti. Li conosce anche il vostro Ministro della salute. Infatti, ha chiesto miseri quattro miliardi, ma non gli date neanche quelli: anzi, gliene togliete. Io non capisco dove volete andare; anzi, forse lo capisco benissimo. Volete smantellare il nostro fiore all'occhiello, la nostra sanità pubblica, che a parole dite tutti di voler difendere e nei fatti distruggete ogni giorno. Si è dovuto scomodare persino il Presidente della Repubblica, che recentemente, proprio nella nostra città, a Torino, ha dichiarato che la sanità pubblica è un bene imprescindibile da difendere - non per niente lo dice anche la nostra Costituzione - e che quindi bisogna mettere più risorse all'interno del Sistema sanitario nazionale: richiamo inascoltato. I nostri medici passano dal sistema sanitario pubblico a quello privato non perché non vogliano lavorare, ma perché li avete messi nelle condizioni di lavorare male; se ne vanno per *burnout*, per esaurimento, perché sono troppo pochi; se ne vanno perché li paghiamo male rispetto all'estero e rispetto alla sanità privata. Penso che ognuno di noi, arrivato a un certo punto, purtroppo prenderebbe delle decisioni. Cosa dobbiamo fare per invertire la rotta, oltre a formare più medici, cosa che, in realtà, abbiamo fatto nella scorsa legislatura? Abbiamo praticamente raddoppiato il numero dei contratti di formazione specialistica per i nostri medici, eliminando quell'imbuto formativo di cui tante volte ci siamo lamentati in quest'Aula. Pertanto, i numeri per sopperire nei prossimi anni al normale *turnover* ci sarebbero - quasi, perché poi rimediare a decenni di mancata formazione non è così facile

pagarli meglio, aumentare gli investimenti e magari fare marcia indietro rispetto a tutte quelle esternalizzazioni che sciaguratamente avete portato avanti per decenni, a partire dai Governi Berlusconi, che - ricordo bene - chiamavano fannulloni i lavoratori del comparto pubblico; salvo poi farli andare a lavorare privatamente, per assicurare profitto agli imprenditori e mal pagare i lavoratori, che si trovano ora al di sotto della soglia di povertà grazie ai vostri provvedimenti. Parliamo di investimenti: si possono fare anche in sanità, come abbiamo detto tante volte. Abbiamo un intergruppo all'interno del Parlamento, che lavora già dalla passata legislatura per far capire a tutti, al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Europa, che anche in sanità si può parlare di investimenti, che non è tutta spesa corrente, spesa infruttifera. Se investiamo

che ci state portando quest'oggi. Sul tema del lavoro, vi riempite la bocca dicendo che il tasso di disoccupazione non è stato mai così basso, ma non spiegate che è basso perché avete precarizzato di nuovo il lavoro, dopo anni di inversione di tendenza. Di nuovo *voucher*, posti a tempo determinato, mentre il numero di contratti a tempo indeterminato cala. Come pensate di porre un freno alla denatalità se la gente non lavora e, quando lavora, è pagata male? Non ci riuscite e si vede dai fatti, perché non volete sentir parlare di salario minimo. Avete anche costretto il CNEL a fare una relazione vergognosa sui possibili danni derivanti tutti i Paesi che l'hanno istituito hanno invece avuto dei benefici. C'è un *mismatch* tra domanda e offerta e c'è un elevato tasso di richiesta, perché per fortuna i cittadini italiani hanno capito che non devono necessariamente fare gli schiavi per qualcuno che li fa lavorare dodici ore al giorno per due euro l'ora.

per la manodopera mal pagata. È per questo che l'avete voluto cancellare, e non certo perché c'erano i fannulloni sul divano. Ma dove stanno questi fannulloni? È il lavoro serio che manca ed è quello che serve nel nostro Paese, quello che voi contrastate perché vi fanno comodo i lavoratori sottopagati e da ricattare. Finisco con l'ultimo richiamo, Presidente - e la ringrazio per il tempo aggiuntivo - sulla sicurezza sul lavoro. Anche in quel caso, tante chiacchiere e pochi fatti. Rafforziamo le agenzie che devono controllare i posti di lavoro; istituiamo la formazione e la cultura della sicurezza nelle scuole e quella procura nazionale del lavoro che tanto ci aiuterebbe per ridurre il numero dei

Paese; riguarda l'aggiornamento delle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, l'aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF e le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo. Secondo quanto esposto dalla NADEF, la manovra di finanza pubblica per il 2024 e il 2026 continua a essere orientata a principi di prudenza, con l'obiettivo di fornire sostegno all'economia attraverso misure mirate ad assicurare il rientro del *deficit* al di sotto del 3 per cento del PIL, in un percorso di riduzione credibile e duraturo del rapporto debito-PIL. Unitamente alla NADEF, il Governo ha trasmesso anche la relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine, ai fini della necessaria

la prima attuazione della riforma fiscale, le misure per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità - quindi rassicuriamo magari anche la senatrice Pirro su questo tema - e il potenziamento degli investimenti pubblici con priorità per quelli previsti dal PNRR e sostegno alle famiglie e alla genitorialità. Voglio ricordare anche che in questi mesi si dovrà discutere sulla *governance* europea. Ricordiamo che che con l'evento del Covid è stata di fatto sospesa la clausola sul Patto di stabilità e dal gennaio 2024, in questa

nelle regole del Patto di stabilità. Ho ascoltato prima i colleghi soprattutto per quanto riguarda il periodo che stiamo attraversando. Non è stato un DEF facile, non è una NADEF facile e non sarà una legge di bilancio facile. Ma credo che la cosa fondamentale in questo momento è essere prudenziali, e quindi ringrazio il ministro Giorgetti per questo. Il ministro Giorgetti si dimostra un buon padre di famiglia, al fine di dare rassicurazione ai nostri cittadini e all'Europa su quanto l'Italia sia responsabile e cerchi di adempiere innanzitutto innanzitutto alle raccomandazioni che derivano prima di tutto dal Consiglio europeo, e quindi sostegno all'economia reale, alle famiglie, alle imprese. il Governo ha investito la maggior parte delle risorse per il contenimento dei costi e anche nella NADEF sono previste risorse per l'azzeramento degli oneri di sistema sulle bollette del gas e la riduzione dell'IVA al 5 per cento sul gas ad uso combustione, teleriscaldamento ed energia,

per l'annualità del 2024 il taglio del cuneo fiscale. Mantenere la liquidità nelle tasche dei dipendenti delle imprese significa dare crescita,

per poter affrontare al meglio l'attuale periodo critico. Ho sentito prima i colleghi parlare di salario minimo. Qui mi sorge spontanea una domanda: perché, se nella scorsa legislatura avevate depositato un disegno di legge su questo tema, avendo una maggioranza, non l'avete approvato? Se eravate così convinti della bontà di questo strumento, per quale motivo non l'avete fatto vostro, ma andate adesso nelle piazze a dire che questa è la misura che tanto serve? Credo che sia stato fondamentale per noi anche far sì che il reddito di cittadinanza esclusivamente alle persone che non possono lavorare. Ancora in questi giorni la CGIA di Mestre ha pubblicato uno studio in cui si parla di una carenza di un milione di lavoratori. Quindi, siccome noi formiamo i nostri ragazzi, cerchiamo di indirizzarli verso professioni per cui possono essere anche *manager*, oppure dei bravi medici. Credo sia importante cercare di fare in modo che queste persone, tramite le politiche

nella legge di bilancio. Forse, se non avessimo fatto 80 miliardi di debito con il superbonus, probabilmente in questo momento avremmo maggiori risorse da poter destinare alle famiglie. Ricordo che quegli 80 miliardi di debito sono serviti per

Sinceramente avremmo tutti sperato, anche soltanto un anno fa, anche rispetto ad alcune indicazioni che abbiamo dato nella scorsa legge di bilancio, di non trovarci in queste condizioni. dell'opposizione o della maggioranza, siamo tutti cittadini di questo Paese: abbiamo le nostre famiglie, gli amici, i parenti, gli elettori. Quando le cose vanno male, nessuno può essere contento; non facciamo come alcuni che pensano di privatizzare gli utili e socializzare le perdite dal punto di vista politico. Quando le cose non vanno non vanno e le cose purtroppo non stanno andando e non solo rispetto all'attualità, cioè quello che stiamo discutendo oggi. Il documento della NADEF, che ci è stato più o meno consegnato un mese fa, è già vecchio rispetto alle emergenze che lo stesso ministro Giorgetti è venuto a illustrarci ieri. Quindi, la situazione - mi dispiace dirlo - non sta per niente navigando e, se oggi Giorgetti dice in manovra di bilancio «tagli duri, saldi diversi se il quadro peggiora», ce la dice lunga. Con onestà intellettuale dobbiamo dire che ci sono dei fatti che non dipendono dal Governo, come le guerre e le le drammatiche notizie di questi giorni, ma ce ne sono altri che noi conoscevamo: l'inflazione, l'incertezza energetica, i temi di cambiamento dello scenario geopolitico e macroeconomico, i tassi della Banca centrale non sono cose misteriose: sono questioni che stiamo analizzando da mesi e, quindi, ci si aspettava una certa NADEF e un disegno dell'economia dei prossimi anni da questo Governo, che è il primo con una maggioranza netta, con un unico progetto politico-culturale che noi abbiamo da anni nel nostro Paese. Questo è stato sbandierato: la prossima legge di bilancio darà darà il segno della nostra visione politica. Questo ci è stato detto da più o meno un anno. E, quindi, ci chiediamo qual è la visione di questa maggioranza politica per i prossimi cinque anni e per i prossimi tre anni nel bilancio, che vedremo poi con quali criteri si farà. È stato detto che questa NADEF è realistica, concreta e prudente.

di crescita. Non è concreta, perché non c'è la visione - e su questo ci ritorneremo - e quindi non ci sono le riforme di cui ho sentito parlare nel dibattito. Non c'è un disegno di concretezza e di pragmatismo sui pilastri di cui questo Paese Paese ha bisogno: penso alla crescita e, quindi, ad azioni anticicliche sulle imprese, sulla produttività. Non c'è nulla, se non in modo peggiorativo, sullo Stato sociale e sui diritti sociali, cioè sulla salute, sull'educazione e sul tema pensionistico.

ribadisco - non dall'opposizione, cioè da enti terzi. Peraltro, ancorare la diminuzione del nostro debito a fantomatiche entrate da privatizzazioni, che non sappiamo quali saranno - e il nostro Paese la dice lunga

La sanità è la grande questione. Oggi si è parlato di sanità e scuola, perché sono due elementi di priorità. Quando le cose vanno male, si sceglie su cosa investire nel medio termine, su ciò che può portare leva al Paese - penso sicuramente al mondo della produzione, quindi innovazione e transizione ecologica

Sulla salute poi c'è di più, perché dopo il Covid tutti abbiamo detto che la sanità italiana sarebbe cambiata e che noi avremmo fatto una scelta di priorità nel Paese per toglierci dalla situazione in cui ci siamo trovati, e cioè rifar ripartire la sanità post-Covid, che non è quella di prima, è un'altra cosa. È stressata, ha il personale sanitario che è stato ridotto allo stremo anche dal punto di vista psicologico, con turnazioni di lavoro e condizioni terribili per più di tre anni, tant'è vero che c'è un abbandono delle professioni sanitarie, da parte non soltanto dei medici, ma anche degli infermieri e dei professionisti sanitari:

modo principale e poi negli altri Paesi. Assistiamo a una fuga del capitale umano. In questo contesto, per la prima volta nei prossimi anni avremo una decrescita del del Fondo sanitario nazionale previsto che passa - come è stato già detto - addirittura al 6,2-6,1 per cento, cioè sotto la soglia indicata dall'OCSE del 6,5 per cento come soglia di sostenibilità dei servizi sanitari. Quando si spende meno del 6,5 del 6,5 per cento rispetto al PIL, crolla il Servizio sanitario nazionale e adesso stiamo tornando a una spesa preventivata nella NADEF, cioè nel disegno, nella visione, che è inferiore. In questo quadro, il prossimo anno, per la prima volta - non è mai accaduto, neanche durante le fasi più difficili della crisi economica dal 2012 al 2017 - abbiamo anche una decrescita in termini assoluti, cioè il prossimo anno

Sarebbero più o meno 4 miliardi. Magari! Ma con quei 4 miliardi che ci facciamo? Quei 4 miliardi coprono l'inflazione. Non c'è nulla di strutturale, non agiamo sul personale sanitario, sulle grandi questioni dell'attrattività, sulle liste di attesa, sui livelli essenziali di assistenza, sulle diseguaglianze tra Nord e Sud, sull'accesso alle prestazioni, sulla medicina del territorio, cioè sulle grandi riforme riforme di cui ha bisogno questo Paese. E non mi venite a dire che non si è intervenuti nel passato, non mi interessa. Ognuno si assume le proprie responsabilità. Oggi c'è il presente e questo presente richiede una presa di consapevolezza comune sul fatto che il combinato disposto della NADEF, della prossima legge di bilancio, dell'autonomia disegnata in modo scellerato da questo Governo, dove non sappiamo neanche cosa succederà dei livelli

seduta con voi per spiegare alla popolazione e creare il consenso per delle scelte che ci permettano di salvare la sanità pubblica in Italia, perché così non andiamo da alcuna parte. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, la Nota di aggiornamento al DEF che oggi ci accingiamo a discutere rivede le previsioni economico-finanziarie non - come è stato poc'anzi detto - in maniera irresponsabile, bensì con prudenza, con serietà e in modo assolutamente realistico, senza i giochi di prestigio o gli effetti ottici

i fattori che hanno determinato il contenuto di questo documento, fattori per lo più negativi o aleatori, sia interni che esterni. Partiamo dai primi, quelli interni, che in qualche modo fanno più rabbia perché erano assolutamente evitabili se solo si fossero applicate dinamiche di buon senso, quelle che avrebbe utilizzato qualunque buon padre di famiglia. Lo ripeto anch'io, riferendomi al superbonus, che solo qualche giorno fa è stato definito una follia da Tito Boeri, l'ex presidente dell'INPS, e che, a conti fatti, riesce a fare ancora peggio delle previsioni. La revisione al rialzo dell'impatto di bilancio dei crediti di imposta legati al superbonus - più 1,1 per causa un conseguente aumento dell'indebitamento netto tendenziale previsto per quest'anno, dal 4,5 al 5,2 per con ben 15 miliardi di euro di scostamento di bilancio necessari a coprire, di competenza e di cassa, la voragine che è stata generata dal cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle. È stata un'autentica sciagura finanziaria che non solo ammorba il presente dei nostri conti pubblici, ma ne ha clamorosamente ipotecato il futuro. E allora, se c'è ancora chi lo rivendica con orgoglio, noi ci troviamo invece costretti a intervenire mettendo una pezza gigantesca, con margini di manovra che sono giocoforza ridotti al minimo, con il senso di responsabilità,

Passiamo ora all'altro punto, che è stato ripetuto e analizzato da chi mi ha preceduto: la sanità. Si legge di tagli, di sistema sanitario nazionale destinato al collasso, ma ci chiediamo: si sta forse parlando dei Governi precedenti? Si stanno forse commemorando i tempi in cui la Sinistra ha calpestato e distrutto un'eccellenza nazionale? Due dati su tutti: i 37,5 miliardi di euro tagliati dal 2010 al 2019. Mi dispiace che non siano presenti illustri rappresentanti di quell'epoca. Non lo dico io, lo dice la fondazione GIMBE. E ricordo anche la favola del 7,4 per cento del PIL investito in sanità nel 2020, uno dei tanti miracoli del presidente Conte, dovuto però al crollo del PIL italiano in pandemia del 9 per cento. È un fiume di menzogne a cui rispondiamo, come al solito, con fatti concreti, destinando risorse per per le cosiddette politiche invariate, quali quelle relative ai rinnovi contrattuali della pubblica amministrazione, a partire dalla sanità appunto. E poi i fattori esterni con cui la NADEF in esame deve fare i conti. Brevemente accenno all'indebolimento dell'economia. Il quadro economico internazionale va ovunque deteriorandosi, con un deciso indebolimento della domanda, in realtà strettamente connessa anche all'*export* italiano (pensiamo ad esempio alla Germania). il rischio di tensioni, da un lato occorre monitorare il più possibile il riacuirsi dei prezzi legati all'energia, dall'altro le eventuali restrizioni nelle catene di offerta e approvvigionamento in settori strategici. Per quanto riguarda la politica monetaria e l'inflazione, anche qui la corsa della BCE a rialzi senza sosta dei tassi di interesse, una cura che invece di salvare il malato Europa rischia di ucciderlo. Per l'Italia qualcosa come 14 miliardi di risorse in meno rispetto a un anno fa, a causa dell'ingente debito pubblico, è un problema. Non solo; famiglie strette nella morsa dei mutui a tasso variabile e fuori controllo e aziende compresse in una difficoltà sempre più evidente nell'accedere al credito. Una vera e propria tempesta perfetta per la nostra economia. Il tutto con effetti a oggi insufficienti in tema di riduzione della spinta inflattiva. Proprio in queste ore, peraltro, la Fed preannuncia una pausa dei tassi. Per l'Unione europea allora, a maggior ragione, perseverare in questa corsa solitaria potrebbe rivelarsi esiziale. E poi il conflitto russo-ucraino; abbiamo fatto una scelta di campo che è stata coraggiosa e dovuta. Abbiamo confermato il nostro pieno sostegno e la nostra fiera appartenenza all'Alleanza Nord Atlantica. Lo abbiamo fatto per difendere il diritto e la libertà. *(Applausi)*. Ciò detto, la libertà. *(Applausi)*. Ciò detto, sono evidenti le ripercussioni dirette e indirette sull'Europa e sull'economia mondiale causate dall'aggressione russa, a cui si aggiungono quelle già oggi evidenti legate al fronte israelo-palestinese. E poi la Cina e i BRICS; anche qui non si può tacere un vento nuovo, ovvero la tendenza di Russia e Cina a privilegiare i flussi commerciali all'interno dei cosiddetti BRICS. È chiaro come un'Europa abbagliata dalla globalizzazione abbia perso la propria indipendenza produttiva e ora rischi di pagare pesantemente il grossolano errore di valutazione in parola.

Gli spazi finanziari generati sul 2023 dallo scostamento per 3,2 miliardi, che serviranno per il conguaglio anticipato dell'adeguamento Istat per l'anno 2024, previsto per i trattamenti pensionistici, per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, come abbiamo detto prima, a partire proprio dalla sanità, e per la gestione dei flussi migratori, che saranno pure, come dicono molti, delle risorse, ma hanno dei costi enormi di integrazione. il taglio del cuneo fiscale è stato confermato anche per il 2024, nell'ottica di una strenua difesa del potere di acquisto delle famiglie e della riduzione del costo del lavoro per le imprese. E ancora il potenziamento di azioni volte a calmierare i prezzi, come fatto con il trimestre antinflazione. Rilevo ancora il sostegno alla crescita grazie ad una efficace revisione e realizzazione del PNRR e del Piano REPower EU, alla dismissione di alcuni *asset*, privilegiando investimenti e partecipazione in settori strategici, quali le reti di comunicazione e le filiere di produzione di semiconduttori, pannelli fotovoltaici e batterie per la riconversione dell'automotive. L'impegno a mantenere sotto controllo il *deficit* e a rientrare entro il 2026 all'interno della soglia del 3 La grande e fondamentale sfida della riforma fiscale, con il passaggio dell'Irpef finalmente a tre aliquote e il mantenimento della *flat tax* per le partite IVA e i professionisti con con ricavi ovvero compensi inferiori a 85.000 euro. Una riforma che ridurrà sensibilmente la pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese; il sostegno alle famiglie e alla genitorialità, premiando i nuclei familiari con due o più figli e riformando puntualmente gli strumenti fiscali loro dedicati; gli interventi mirati sul caro energia, riservati a famiglie e imprese in difficoltà. Insomma tanti fattori di criticità, certo, ma anche tanta visione e tanta programmazione; una NADEF che preannuncia una manovra che sarà ancora una volta Anche qui non sono io a dirlo: c'è un'Italia resiliente, straordinariamente resiliente, pure in un contesto che mette a dura prova storici punti punti di riferimento come la Germania. Abbiamo l'orgoglio di richiamare il successo del BTP Valore, con una raccolta di oltre 17 miliardi di euro, e la vitalità del mercato del lavoro, con dati che sono eccezionali rispetto a un anno fa. a un anno fa. Signor Presidente, concludo con un appello. Noi non chiediamo a chi siede dall'altra parte, tra i banchi dell'opposizione, di mettere a posto i danni che loro stessi hanno causato, perché lo stiamo facendo noi, lo fa il Governo Meloni. Una cosa però dovete farla: parlare in modo diverso dell'Italia in Europa e nel mondo. Non si difendono i falsi miti o, peggio, la falsa speranza di poter ribaltare il voto popolare con dei sotterfugi e dei giochi di palazzo. Si smetta di tifare per lo *spread*, per rievocare gli attacchi speculativi della Bundesbank. *(Applausi)*. PRESIDENTE. Grazie, senatrice Ambrogio. È andata due minuti oltre il tempo. Concluda, prego.

vi sembrerà strano, però vorrei iniziare anch'io parlando della sanità. Vorrei iniziare il mio intervento illustrando la situazione nella quale versano i due ospedali della mia Provincia,

L'ospedale di Merate, presidio sanitario fondamentale per il nostro territorio, facendo parte della ASST di Lecco, rispetto al quale ho presentato anche un'interrogazione parlamentare, negli ultimi anni ha registrato una riduzione dei posti letto e dell'attività delle sale operatore. In particolare, poi, la cosa si è accentuata dopo il Covid: si è partiti con le dimissioni del primario di chirurgia, si è ridotto il reparto di psichiatria, si è ridimensionato il reparto di ortopedia, il cui medico primario si è dimesso, e si sono accorpati una serie di reparti, riducendo i posti letto. Il pronto soccorso funziona sostanzialmente con due medici a tempo pieno e uno *part time*, e tutto a gettoni. In sostanza, abbiamo una situazione in cui, ad esempio, le operazioni si riducono di molto, perché il 50 per cento degli anestesisti si è dimesso e quindi le attività operatorie sono ridotte.

ad esempio si sono dimessi quattro oculisti su cinque del reparto di oculistica, tra cui il primario; capite voi stessi qual è la situazione. In più sono successi due fatti, proprio la settimana scorsa. Nel reparto di chirurgia si sono presentati diciannove pazienti, ma c'erano solo tre posti letto e li hanno rimandati indietro. Il giorno successivo in ginecologia si sono presentate quattro partorienti e il medico ha detto loro: c'è un solo posto, decidete voi chi rimane. Siamo in questa situazione non nel paese più sperduto d'Italia, ma a Lecco, una delle città che ha il reddito più alto di questo nostro Paese. Quindi, la situazione è questa.

Si fa questa scelta perché la destra, voi che state governando, come avete sempre dimostrato nella mia Regione, cioè in Lombardia, privilegiate il privato rispetto al pubblico. pubblico. La sanità pubblica universale, che deve rispondere alle esigenze dei cittadini, praticamente viene messa in discussione. Le chiacchiere non servono.

che intervenga sulla costruzione di case popolari, sul ripristino delle case popolare, che ci sono, sulla messa in sicurezza delle case popolari, che ci sono. Intervenire sul mercato, come si usa dire, visto che

Le dice il fatto che, ad esempio, una confederazione come la Confesercenti ci dice che si preannuncia un autunno freddo per le famiglie e le imprese. Quindi, in sostanza, questa NADEF non

bisogna affrontare oggi il problema di chi lavora, quindi forse l'immigrazione va affrontata con un altro piglio e con un'idea diversa di integrazione in questa società. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paita. Ne ha facoltà. Signor Presidente, all'inizio di questo mio breve ragionamento vorrei fare un tuffo indietro, come se il ritorno al futuro potesse essere ancora una metafora utilizzata Voglio ricordarmi le ragioni e gli argomenti con i quali questo Governo e le forze politiche che appartengono a questo Governo hanno affrontato la campagna elettorale. Tra quelle ragioni - spero di non dimenticare i temi più importanti - c'era: la grande questione della lotta all'immigrazione, addirittura con l'ipotesi del blocco degli sbarchi e quindi con un Governo che aveva in mente una strategia di riduzione dei flussi verso il nostro Paese; il tema della lotta alle tasse, quindi una diminuzione consistente del livello di tassazione nel nostro Paese; della cosiddetta legge Fornero, che doveva essere immediatamente messa in campo al fine di rivedere il tema del sistema pensionistico. Non mi esprimo su quello che penso di queste tre strategie perché è noto a tutti; dico solo che di queste tre strategie non è rimasto nulla: i migranti nel nostro Paese sono aumentati, anzi sono triplicati; della riforma delle pensioni non c'è traccia alcuna; alcuna; le tasse stanno aumentando. Assieme a questo, voglio ricordare che abbiamo un *deficit* che sale nel 2023; abbiamo il PIL che crescerà dell'1,2 per cento, ma è una stima al ribasso rispetto alla stima fissata ad aprile dell'1,5 per cento; abbiamo un debito che continua ad essere del

è l'Ufficio parlamentare di bilancio a dire che le prospettive economiche, in particolare quelle sull'indebitamento, sono tutt'altro che rassicuranti. Non sono io, ma sono i numeri a identificare in questa NADEF una prospettiva di taglio del *welfare* e un'incapacità reale di produrre investimento. È una regola: è chiaro che se tu non cresci, redistribuire è difficile. Questo scenario naturalmente mitiga il ragionamento che sto facendo alla luce di quello che sta avvenendo attorno a noi (nessuno è chiuso nel proprio orticello), ma è chiaro che dal punto di vista della capacità di crescere di questo Governo siamo di fronte a problemi grossi e chi vi parla non è espressione di una forza politica che tifa lo *spread*. Noi tifiamo per il Paese, tifiamo per il Paese sempre e alla luce del nostro atteggiamento sempre responsabile, sempre nel merito, possiamo forse, anche più credibilmente di altri (che magari, quando possono, fanno pure il tifo perché le cose vadano male), dirvi che ci sono dei problemi e che mettere la testa sotto il tappeto non aiuterà a risolvere il problema dell'Italia: non calmerà i mercati, non aiuterà ad affrontare il tema dello *spread* e non aiuterà ad affrontare il nodo di quella crescita modesta della quale parlavo prima. Vi cito un esempio, perché, per quanto mi riguarda e per la mia formazione politica, questo è uno dei temi più importanti: la politica industriale. Mi spiegate chi sta facendo la politica industriale in questo Governo? *(Applausi)*. Chi si sta occupando di questioni fondamentali come il tema dell'Ilva? Parliamo di un'enormità di lavoratori che sono in cassa integrazione, parliamo di impianti che dovevano avere un ammodernamento e che sono stati lasciati lì. Parliamo di un Governo che balbetta e in particolare a farlo è il ministro

il tema dell'acciaio è collaterale e fondamentale a tutto il resto del sistema produttivo. È inutile parlare di grandi questioni, è inutile parlare dell'*automotive,* se poi non si affronta questo tema in maniera seria. Chi vi parla è cittadina di una Regione dove il ruolo dell'Ilva è stato importantissimo, ma non dimentico anche l'apporto di Taranto a questo tipo di causa e a questo valore dal punto di vista della produzione nazionale. Chi si sta occupando dei temi industriali? Perché io sento parlare di tutto, sento parlare ogni giorno di un decreto nuovo che darà una stretta giuridica, che produrrà risultati in termini di legalità fantasmagorici, ma una parola sulle questioni industriali del nostro Paese questo Governo non la sa dire. Poi c'è un'altra questione (mi limito ovviamente a due, tre grandi temi per ragioni di tempo): nella NADEF si prospetta un taglio ulteriore al Servizio sanitario nazionale. Qui siamo in una sfera che è una vera e propria emergenza, perché se sommiamo inflazione, aumento dei tassi e ulteriore taglio alla sanità, si ha di fronte la prospettiva di un cittadino italiano che (altro che aiutare i più deboli) deve scegliere se mangiare o curarsi. Questo, dal mio punto di vista, è l'aspetto più drammatico, perché se devo affrontare liste d'attesa inaccettabili e non ho la possibilità di ricorrere al privato per fare esami diagnostici, significa che la mia prospettiva di vita, in in relazione alla mia collocazione e appartenenza sociale, subisce un cambiamento. Penso a genitori che magari devono curare i propri figli, penso a persone che non sono in grado di affrontare quelle liste di attesa. Guardate che è inutile dire: basta che tutti i cittadini vadano al pronto soccorso. Per non andare ai pronto soccorso ci vuole una rete di servizi adeguati, ci vuole una capacità sul territorio di ridisegnare il sistema sanitario e voi non solo state ridisegnando il sistema sanitario, ma state tagliando quello che c'è o prospettate di farlo. Ho sentito il ministro Giorgetti, verso il quale nutro stima, perché è una persona seria, ma lui si è un po' arrampicato sugli specchi anche in Commissione su questo punto, perché non ha il coraggio di dire che quello è lo scenario e non è in grado di dire se nella legge di bilancio quel taglio ci sarà oppure no. Allora, su questo punto faccio un appello anche ai colleghi della maggioranza. Il tema della sanità è cruciale per il nostro Paese, non solo per difendere un sistema sanitario che ha dato risposte a tanti cittadini,

tecniche, ma sono profonde, profondissime ragioni politiche che ci portano a dire che, a un anno dal vostro insediamento, i problemi di questo Paese non sono diminuiti, ma di molto aumentati.

che con i se e con i ma non si fa la storia, ma è evidente che in condizioni mondiali differenti oggi avremmo avuto dei margini di azione molto differenti, molto più ampi per questo

che servono per fare una manovra finanziaria e per realizzare tante di quelle cose che anche le opposizioni oggi ci chiedono e che noi facciamo e faremo con la manovra di bilancio di qui a breve. 23,5 miliardi, 3 miliardi serviranno per l'indicizzazione delle pensioni, per un miglioramento dei contratti di lavoro e anche per la sanità, da utilizzare subito, come gli altri 20, per poter dare attuazione anche a tutta una serie di riforme che abbiamo messo in campo, per intervenire sul

Le nostre parole d'ordine sono crescita e occupazione ed è su questa linea che il Governo si è sempre mosso e si sta muovendo. Questa è la strategia e i risultati arrivano, perché il tasso di disoccupazione oggi scende e quindi siamo ancora impegnati su certe misure importanti che servono a farlo scendere

anche con gli investimenti ed ecco perché siamo impegnati fortemente nella piena attuazione degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che sono importanti per la crescita del nostro Paese. La riforma fiscale, che da pilastro sostenuto e voluto da Forza Italia e dal centrodestra, finalmente può vedere, grazie a questa manovra finanziaria, la riduzione degli scaglioni a tre, consentendoci di continuare su quelle politiche di *flat tax* per partite IVA e professionisti. Questi sono gli obiettivi che il Governo si è dato e che sta raggiungendo in una visione complessiva, in uno scenario internazionale difficile, soprattutto in una prospettiva di legislatura. È su questo che è importante oggi lavorare: sulla stabilità. Molti nell'opposizione ci vogliono divisi e separati, invece questa

positive che sono state fatte in questi mesi, perché l'economia italiana è solida, ha dei punti di forza importanti sui quali fare leva, come la competitività internazionale e un settore finanziario solido. quindi delle caratteristiche necessarie oggi per puntare allo sviluppo. Il Governo opera in uno scenario difficile, sta facendo passi in avanti importanti nonostante le grandi difficoltà

degli italiani e del nostro Paese. Lo farà anche con la legge di bilancio, che varerà nelle prossime settimane e siamo sicuri e convinti che, se anche ci sarà un momento difficile di restrizione, come sempre noi saremo qui in Parlamento a sostenerlo e con le misure che oggi gli italiani ci chiedono.

la NADEF che ci apprestiamo a votare delinea un quadro desolante rispetto alla prossima legge di bilancio, con prospettive troppo ottimistiche, così come è stato evidenziato nelle audizioni della Banca d'Italia, d'Italia, dell'Ufficio parlamentare di bilancio e della Corte dei conti, e rischia di essere un vero e proprio libro dei sogni in relazione anche alle prospettive poco realistiche di legge di bilancio si preannuncia peraltro senza margini di crescita, poco ambizioso, senza una visione - nonostante dopo tanti anni l'Italia abbia un Governo politico - basato sul debito, sui tagli e sulle privatizzazioni. La NADEF dimostra anche tutta l'incapacità del Governo, che non ha creato i presupposti della crescita, non ha realizzato una politica degli investimenti, non ha realizzato riforme strutturali utili al Paese e, soprattutto, non ha rispettato le scadenze di spesa del Piano nazionale di ripresa resilienza. basta, infatti, una norma, non basta accentrare i poteri; occorre governare i processi di spesa. È lì che si misura la capacità e la professionalità di un Governo. Noi abbiamo lasciato una locomotiva, peraltro la più veloce d'Europa. Adesso ci troviamo con un Paese fermo,

Avete previsto una crescita dell'1,2 per cento, ma avete dimenticato forse di analizzare i risultati del secondo e terzo trimestre, negativi, dell'anno in corso. Avete dimenticato quali sono le previsioni dei risultati della seconda metà dell'anno in corso e avete anche dimenticato quali sono i rischi all'orizzonte: consumi in calo, tassi di interesse elevati, uno *spread* che dà già segnali di forte preoccupazione e, soprattutto, il risveglio dei prezzi - in aumento - del petrolio e del gas ed una inflazione che rischia di rimanere sopra il 5 per cento. La legge di bilancio muoverà 25 miliardi a fronte di una crescita quasi nulla. Crescere dello zero virgola significa infatti crescita nulla. Sapete qual è l'impatto di questi 25 miliardi sulla crescita incrementale? Solo dello 0,2 per cento, quindi nulla. Questo però dimostra una cosa: dimostra che tutte le misure che voi andrete a varare e che avete quindi già programmato non solo sono inefficaci e le risorse che andrete a stanziare sono insufficienti.

non punteranno a quella crescita che ci permetterebbe di coprire l'onerosità di questo maggiore debito, per cui il rischio è tornare indietro al 2010, quando il Paese è entrato nella cosiddetta trappola del debito. Oltre 40 miliardi di incremento degli interessi passivi che non saranno coperti da quello 0,2 per cento. Sapete qual è il rischio? Il rischio è una voragine nei conti pubblici. State creando un buco nell'acqua e le preoccupazioni di Banca d'Italia, della Corte dei conti e dell'Ufficio parlamentare di bilancio vi chiedono di correggere e di valutare meglio i conti. Cosa facciamo, cosa fate, anzi, con lo scostamento di bilancio? Poche cose. Un taglio del cuneo fiscale, che confermate, senza renderlo peraltro strutturale; estendete poi il primo scaglione Irpef

state solo dando un contentino ai redditi più alti. Attenzione, però, non vi siete dimenticati le spese militari, che aumenteranno: è l'unica voce che aumenterà in questo nella prossima legge di bilancio. *(Applausi)*. Vi elenco le cose che invece non fate. Non sostenete un piano sugli investimenti, tagliate la spesa pubblica alla scuola e alla ricerca, non adeguate e non aumentate i salari e le pensioni del ceto medio.

che chiediamo al Parlamento di votare e di approvare una legge sul salario minimo legale, ma non abbiamo avuto i numeri per poterlo fare, perché eravamo l'unica forza politica. Adesso siamo contenti che anche le attuali forze di opposizione si siano accodate e stiano sostenendo quest'azione di civiltà. Vi siete dimenticati altresì della povertà, dell'inflazione, del caro mutui e del caro affitti. Attenzione, però: c'è un grande *bluff* in questa legge di bilancio, con il mancato superamento della legge Fornero, che avevate promesso; una riforma fiscale in cui avevate annunciato un ampliamento della *flat tax*, che non riuscirete a fare; una detassazione delle tredicesime che avete annunciato, anche in pompa magna, ma che non ci sarà nella prossima legge di bilancio. L'inutilità di questo scostamento è inoltre attestata anche dal fatto che non riducete il debito pubblico, che si cristallizzerà al 140 per cento. Dato che si parla sempre di superbonus e di indebitamento, che anche quando noi abbiamo governato questo Paese, in piena pandemia, i soldi non c'erano: noi siamo andati a trovarli e li abbiamo spesi (parlo di oltre 150 miliardi). Sapete di quanto è stata la riduzione del debito pubblico? Di ben 14 punti base.

ma avete letto e studiato la storia economica degli ultimi anni? Quando mai lo Stato italiano ha realizzato in così poco tempo una privatizzazione di tale portata? 20 miliardi: mai accaduto. Abbiamo la preoccupazione che queste privatizzazioni non si realizzeranno e ci sarà un vero e proprio buco di bilancio: altro che il superbonus. *(Applausi)*. Abbiamo poi la revisione della spesa. Non sappiamo cosa andrete a tagliare.

Evasione fiscale, contrasto all'evasione fiscale e taglio ai sussidi ambientali: 30 miliardi, subito. Concludo, Presidente, con una citazione del professor Soriano («L'inconveniente umano»). Il vostro Governo assomiglia a certi temporali estivi: fanno un gran baccano, durano poco e spesso - anzi, in e spesso - anzi, in questo caso, ne abbiamo la certezza - si lasciano dietro un grande danno. Signor Presidente, Governo, colleghi, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza si sviluppa nella logica del concetto della prudenza, della concretezza e della schiettezza nella relazione Stato-cittadino, consolidando l'orizzonte di crescita del PIL mediante azioni che rendano più competitivo il nostro Paese, soprattutto verso quei mercati che negli ultimi tempi hanno manifestato qualche cedimento nell'importazione dei nostri prodotti (mi riferisco a Francia, Germania, Stati Uniti), pur avendone grandi potenzialità, per poi assicurare la finalizzazione di risorse, nonostante il periodo congiunturale, e dovendosi evitare che si continui a generare debito senza prima aver percorso la strada della razionalizzazione e aver misurato gli effettivi fabbisogni. Io mi soffermerò solo sul capitolo sanità. Ebbene, il nostro apprezzamento al documento in esame è dovuto all'oculatezza dei passi che si intendono intraprendere, perché, data la relatività delle risorse disponibili, frutto delle criticità cristallizzate nel tempo, prima fra tutte l'aumento del costo per interessi dovuto al debito *monstre*, con esborsi superiori ai 100 miliardi su base annua, sono state previste importanti direttrici di sviluppo e relative misure correttive, con risorse senz'altro inadeguate rispetto ai bisogni, a cominciare proprio dalla sanità, ma con la consapevolezza di aver fatto al momento il possibile e di fare ancor di più in manovra di bilancio, con ulteriori incrementi per consolidare sul 2024 più di quanto stanziato quest'anno, in modo da proiettarsi sul triennio verso l'obiettivo tendenziale dei 140 miliardi. La NADEF dà infatti contezza di una spesa sanitaria che ha crescenti necessità statistico-epidemiologiche di essere rivista al rialzo. È da qui che nasce l'esigenza di trovare soluzioni più performanti, in grado di dare di più e costare di meno (lo ripeterò), riducendo le disomogeneità, ma nel contempo incitando coloro che sono stati meno performanti a saltare qualche passaggio tecnologico, in modo da essere celermente alla pari rispetto agli *standard* minimi dei livelli essenziali delle prestazioni cui debbono tendere i nuovi LEA. Tutto questo in un approccio effettivamente integrato ospedale-territorio, marginalizzando le inappropriatezze sia in prevenzione sia in cura, con nuove e innovative regole di ingaggio di tutti gli erogatori e di contrattualizzazione dei professionisti per minimizzare le liste d'attesa, ricorrendo all'innovazione, alla digitalizzazione e alla telemedicina, con revisione aggiornata dei DRG e delle tariffe secondo il principio del giusto corrispettivo, sulla base dell'analisi dei costi, del valore clinico e dei prezzi, con incisivi, stringenti meccanismi di valutazione e controllo. Programmazione, valutazione e controlli sostanziali: dunque nel solco delle direttrici ordinamentali dei disegni di legge che abbiamo promosso per il riordino dell'emergenza-urgenza e il potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria, ma non mi pare che tra di noi ci sia qualcuno in grado di fare magie, d'altronde l'università di Exeter ha introdotto solo quest'anno i relativi corsi e chi ha annunciato sovrabbondanza di risorse per dispensare sussidi e *bonus* illimitati, quand'anche in buona fede, sperando di generare un volano motore, ci ha lasciato un conto da 130 miliardi di euro. *(Applausi)*. Situazione sicuramente unica, ma unico anche il conto.

anche un intervento legislativo in materia di riordino, riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale e dell'assistenza ospedaliera nel Servizio sanitario nazionale. Difatti, al riguardo, dobbiamo avere contezza che, a risorse date, con il PNRR upgradato si possono fare molti interventi progettuali moltiplicatori di PIL, unico fattore in grado di permettere un incremento di risorse in sanità, ma il loro funzionamento gestionale dipende essenzialmente dalla capacità di fare *saving* ragionato, riallocando e riqualificando risorse umane e prestazionali sulla base dei bisogni. Ora, per arrivare a una sanità davvero equiaccessibile, universalistica e sostenibile nel tempo, non smetto mai di sottolineare quanto ne sia precondizione disporre di medici e operatori molto preparati, su cui occorre investire quantitativamente con competenze digitali avanzate, ma non basta. Occorre una visione d'insieme, che sin qui è stata poco applicata, una visione strategica complessiva che si snoda attraverso interventi e misure non solo congiunturali, ma di carattere ordinamentale, propedeutiche al cambiamento necessario. Ed è per questo che sono necessari interventi, come dicevo, normo-ordinamentali che incidano significativamente nell'orizzonte del cambiamento necessario, anche in materia di medicina difensiva, integrando prevenzione, emergenza-urgenza e medicina territoriale in chiave di sostenibilità nel medio-lungo periodo, a garanzia di continuità e di tempestività delle cure, anche in elezione, contrastando incongruenze e disfunzioni non più sostenibili in tempi di crisi, dunque

che contribuirà in modo significativo a liberare risorse per la normalizzazione dei tempi d'attesa con CUP integrati, senza accampare ulteriori scuse dilatorie nella trasparenza delle agende pubblico-privato, evitando le pratiche inappropriate per dare di più costando di meno, dovendosi percorrere strade diverse da quelle che i problemi li hanno generati. Signor Presidente, mi avvio Se i primi provvedimenti possono considerarsi relativamente semplici, quanto più ci si avvicina all'obiettivo dell'efficienza, maggiore

per noi la NADEF rappresenta un passaggio politico importante; per noi non è un esercizio di esclusiva competenza degli economisti. signor Presidente, di essere rimasto molto sorpreso ieri dalla scelta del Governo in Commissione bilancio di rinunciare alle repliche dopo la discussione generale. Soprattutto, anche la scelta del Presidente di procedere al voto senza i pareri delle Commissioni parlamentari più importanti non è un fatto tecnico,

invece un alto valore politico, perché la politica economica definisce l'identità di un Governo: racchiude valori, oltre a definire la legislazione vigente e la cornice entro la quale si muoverà la legge di bilancio, quindi non siamo in presenza di un fatto tecnico, poiché è una grande questione politica quella che dobbiamo affrontare; soprattutto se vogliamo restituire alla politica il ruolo che la Costituzione ci assegna, non possiamo ignorare questi passaggi. Lo dico subito in premessa: noi non neghiamo e non ignoriamo il difficile contesto economico all'interno del quale si muovono i saldi di finanza pubblica e l'iniziativa del Governo. Siamo in presenza di un rallentamento dell'economia mondiale, anche a causa delle politiche monetarie restrittive, è un dato di fatto. A nostro avviso, non era perché dopo un ciclo lungo di inflazione le banche centrali rialzano i tassi. Se aggiungiamo a tutto questo il contesto e il tumulto che esistono in Europa con la guerra in Ucraina e oggi in Medio Oriente, ci rendiamo perfettamente conto che la fase alla quale andremo incontro richiede qualità dei Governi, ma soprattutto azioni riformatrici vere e autentiche sui pilastri strutturali dei limiti e delle difficoltà economiche e sociali di questo Paese. Nel secondo trimestre, il PIL si è ridotto dello 0,4 per cento rispetto al periodo precedente (parliamo del 2023), all'interno di una fase ciclica certamente debole, ma la narrazione di questo Governo, questi mesi, è sempre stata orientata a determinare un'immagine del nostro Paese quasi che ci trovassimo all'interno di un *boom* economico, quasi che potessimo scamparla dai problemi strutturali che invece attraversano anche la crescita europea. Questi sono i dati. sono i dati. Aggiungiamo la fine della sospensione del Patto di stabilità e l'avvio di un nuovo ciclo di programmazione europea al costo del debito che nei prossimi anni arriverà a 104 miliardi di euro. oggi invece siete qui a chiedere a questo Parlamento in *deficit* un'autorizzazione senza alcuna finalizzazione, senza una visione, senza un progetto per lo sviluppo economico di questo Paese. Non c'è un'idea su come fare crescere questo Paese. Non c'è uno straccio di proposta in una programmazione triennale, certo a legislazione vigente; aspetteremo la legge di bilancio, sperando che ci porti il miracolo voi fin qui avete a parole enunciato, ma nei fatti negato e contraddetto. Sappiamo tutti, non c'è bisogno di tante lauree in economia, che il sentiero per sostenere il debito è una nuova crescita economica. Ascoltando i vostri interventi - lo voglio dire fin da subito - l'unica cifra che emerge dalle vostre considerazioni è la retorica di un'opposizione al passato. al passato. Lo vogliamo dire con grande chiarezza: l'esercizio dell'opposizione al passato può funzionare per costruire un consenso di breve termine nel rapporto con il Paese, perché spesso è utilizzata da voi per nascondere le vostre lacune, ma guardate che non produce niente per le giovani generazioni e per il futuro di questo Paese. È un perder tempo in un'opposizione al passato. Se dobbiamo leggere il passato, usciamo da una fase pandemica ed entriamo in un nuovo ciclo di programmazione economica europea e dobbiamo prendere in mano il terreno dello sviluppo economico, della trasformazione di limiti strutturali che in questo Paese insistono. Cominciamo a vederli, a leggerli: per poter affrontare questo processo di innovazione economica, dovete credere nella trasformazione in chiave ecologica dell'economia come fattore di competitività e non come rischio per l'occupazione, per il disagio e per il lavoro. Noi vogliamo portare all'interno del cambiamento in atto le condizioni economiche ed ambientali: le questioni ambientali devono diventare per voi la priorità, se vogliamo costruire nuovo sviluppo economico, e non possono essere negate. Voi siete al negazionismo delle trasformazioni. *(Applausi)*, non a nuove politiche economiche: questo capita sia nelle dinamiche dei processi di digitalizzazione, sia nelle dinamiche sociali. Una fase così complessa richiederebbe un piano straordinario di riforme, Presidente, e non l'utilizzo delle riforme come arma di distrazione di massa: voi volete piegare questo Paese a discutere di presidenzialismo e volete costringere questo Parlamento ad affrontare il tema dell'autonomia differenziata in quanto collegato alla legge di bilancio, senza oneri per la finanza pubblica, pensando che queste riforme producano un contributo alla crescita? Per me dovete cambiare strada. Le vere questioni che dobbiamo affrontare sono altre, per il Partito Democratico sono chiare e ve le vogliamo dire, perché non si dica mai che non abbiamo proposte. Prima questione: in questo Paese continuiamo a pensare che il lavoro debba e possa essere sottopagato e indegno, siamo pieni di precarietà e dunque mangiamo futuro a questo Paese con la crescita della precarietà e del disagio sociale, per cui le giovani generazioni perdono la speranza di competere nella qualità della vita di questo Paese. Ecco perché dovreste non usare il CNEL come arma di distrazione di massa per affossare il salario minimo, ma affrontare voi la questione salariale come fattore di competitività *(Applausi)*, se volete essere un Governo serio che guarda alle generazioni e non sempre alla costruzione populistica e propagandistica del consenso per le elezioni. Seconda questione, altrettanto importante, dopo quella salariale, che per noi è fondamentale, perché restituire dignità alla parola lavoro vuol dire aprire un sentiero nuovo di speranza e di competitività economica.

invece di praticare la lotta all'evasione e di salvaguardare il principio di progressività nel sistema fiscale,

l'innalzamento del tetto all'utilizzo del contante, l'abbandono e la messa da parte dei processi di fatturazione elettronica, di digitalizzazione, di tracciabilità dei pagamenti. Noi vi chiediamo da subito di portare finalmente in quest'Aula un'analisi puntuale su come stanno andando le entrate fiscali e su cosa sta producendo il messaggio ambiguo, sbagliato e profondamente iniquo, cui il sistema fiscale italiano è un peso. Dobbiamo ristabilire un patto di fedeltà fiscale e dunque, al posto dell'autonomia differenziata, serve la riforma del Sistema sanitario nazionale. Perché non individuate le priorità di cui il Paese ha bisogno? Oggi un lavoratore dipendente è costretto a pagarsi le prestazioni sanitarie sanitarie e a spendere risorse importanti, che sottrae dai consumi interni, per potersi curare. Abbiamo bisogno di una riforma urgente del sistema sanitario, oltre che delle risorse necessarie per ricalibrare il rapporto tra spesa sanitaria e prodotto interno lordo che voi avete profondamente ignorato. Ignorare questo fenomeno vuol dire rompere in profondità il tessuto sociale e culturale che costituisce nella fedeltà fiscale un patto tra cittadino e Stato. Non è un danno alla destra quello che vi stiamo chiedendo. Voi state facendo un danno al Paese. Togliete di mezzo le tre parole che state utilizzando. Questa non è una cornice di bilancio ispirata ai princìpi della della responsabilità, della realtà e della prudenza. Non è prudente, signor Presidente, sovrastimare la crescita, individuare un punto di PIL sulle privatizzazioni senza indicare alcuna strada. Non è prudente continuare a favorire l'evasione, anziché qualificare un grande progetto di crescita economica e di sviluppo del Paese.

con pragmatismo e grande responsabilità. Il rallentamento del quadro macroeconomico registrato negli ultimi mesi, il deterioramento delle prospettive di crescita a livello globale e una dinamica dei prezzi ancora sostenuta incidono sensibilmente sul potere di acquisto delle famiglie e sulla competitività delle nostre imprese. Dopo il 2021 e il 2022 l'economia italiana ha recuperato rispetto alla caduta del 2020, ma ancora in modo troppo debole. A livello congiunturale questi segnali si sono tradotti in una riduzione del PIL pari a quattro decimi di punto nel secondo semestre. Pur in un quadro non facile, il mercato del lavoro ha risposto e dobbiamo ricordare che quest'anno (proprio quest'estate) c'è stato il *record* di occupati nel sistema Italia dal 2004 ad oggi. E questo è un grande successo del Governo Meloni in una congiuntura non facile. L'Italia che produce e che crea ricchezza e posti di lavoro non si è mai arresa, nemmeno di fronte alle difficoltà. Il rallentamento in atto è spiegato da una incertezza e da un quadro internazionale di riferimento molto difficile, segnato da un calo della domanda globale e da un inasprimento delle condizioni monetarie e finanziarie.

Purtroppo - a mio a mio modo di vedere - la Banca centrale europea sta seguendo in modo troppo pedissequo quello che sta facendo la Fed negli Stati Uniti.

interna, c'è una grave crisi economica interna e non è un caso che la Fed stia stampando *trillion* di dollari per sostenere le imprese americane. L'inflazione che abbiamo oggi in Europa è, invece, esogena, causata da fattori esterni, dalla guerra in Ucraina all'aumento delle materie prime, all'aumento dei costi delle merci.

mentre negli Stati Uniti oltre il 90 per cento degli investimenti e dei mutui delle imprese è a tasso fisso, in Europa è l'esatto opposto. Quindi, l'aumento dei tassi in Europa ha creato gravi problemi alle famiglie e alle imprese. Per quanto riguarda l'inflazione, se dobbiamo dirla tutta, c'è anche un fattore endogeno,

Incombe anche il rischio, a livello geopolitico, di un acuirsi delle tensioni internazionali. Purtroppo è di questi giorni il verificarsi di gravissimi fatti in Medio Oriente, dove Israele è fatta oggetto di un attacco criminale crea ripercussioni in gran parte del Mediterraneo. Sono situazioni che potrebbero dare luogo a nuovi *shock* ai prezzi dell'energia. Alla luce della crescita leggermente al di sotto delle aspettative dell'attività economica prefigurata per il secondo semestre, tali fattori portano a ritoccare le stime che il DEF aveva posto all'uno per cento, che oggi vengono ritoccate allo 0,8 Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione e del fabbisogno di cassa del settore pubblico dell'anno scorso hanno fortemente risentito dell'impatto di crediti di imposta (superbonus) legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia. In particolar modo il superbonus - come ho detto prima - era un buon provvedimento, ma scritto male e finito peggio. La strategia del Governo si basa dunque sulla individuazione di un punto di equilibrio tra sostegno alla crescita, agli investimenti e al potere d'acquisto delle famiglie italiane - da un lato - e disciplina di bilancio e riduzione del rapporto debito-PIL, dall'altro. Ciò sarà possibile anche attraverso dismissioni di partecipazioni societarie pubbliche, rispetto alle quali esistono impegni nei confronti della Commissione europea legati alla disciplina sugli aiuti di Stato. Questo è un Governo responsabile, consapevole, coerente e pragmatico, conscio che la rotta da seguire e mantenere è quella della sostenibilità di un debito pubblico molto elevato. lo Stato, grazie al Governo Meloni, passa da uno Stato assistenziale a protagonista nello scenario della politica industriale. Qualcuno

vorrei dire alla collega Paita che oggi abbiamo uno Stato stratega, uno Stato che vuole fare gli interessi della Nazione. Non è un caso che il *golden power*, per il quale abbiamo votato qualche mese fa, sia uno strumento che lo Stato utilizza proprio da un punto di vista strategico. Qualcuno ha detto che è stato utilizzato molte volte.

consigli, di provvedimenti che cercavano di dare un indirizzo a chi doveva fare determinate acquisizioni. Quindi lo Stato, quando interviene, oggi, lo fa nell'interesse nazionale e non perché vuole fare una politica di programmazione sovietica come qualcuno vuole far intendere. Parliamo ora di sanità, e prima la collega Ambrogio l'ha ricordato. La fondazione GIMBE dice che dal 2010 al 2019 i Governi hanno tagliato 37,5 miliardi alla sanità.

riparto pensando che l'Italia sia più forte, ora più di quanto non fosse un anno fa, e non si può dire lo stesso degli altri sistemi economici europei, quindi avete un motivo in più per essere ottimisti. Il Governo Meloni? Si è dimostrato più forte del previsto. Sono pronto a co-investire con aziende italiane sulle infrastrutture della vostra Nazione.

caro collega Turco che prima citava il professor Saviano che parlava del Governo come di un temporale

oggi la stabilità del Governo Meloni e la sua prospettiva temporale stanno diventando un'attrattiva per questo tipo di fondi che guardano a realtà stabili e in crescita.

dai senatori Malan, Romeo, Ronzulli e Biancofiore. Sono inoltre pervenute alla Presidenza, sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023,

sono in distribuzione.

sulla proposta di risoluzione presentata alla relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, nonché di indicare quale proposta di risoluzione relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza intende accettare.

NADEF è molto realistica ed è scritta in un quadro economico e geopolitico globale caratterizzato da elevata volatilità, come testimoniato in queste ore dal drammatico riacuirsi del conflitto israelo-palestinese, oggetto della nostra seduta d'Aula ieri, o ancora dall'elevata inflazione mondiale. mondiale. Noi non siamo fortunati: l'inflazione non ci fa beneficiare nemmeno dell'effetto del calo dei prodotti energetici, perché - come abbiamo dovuto apprendere proprio ieri - a causa della guerra in Israele purtroppo questi continueranno a pesare sui conti pubblici e sulle tasche degli italiani, quanto la permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, aggravata appunto da quella in Medio Oriente. In aggiunta, la sostanziale stagnazione dell'economia europea e la contrazione del commercio mondiale nel secondo trimestre di quest'anno hanno inevitabilmente causato una temporanea e - si spera - lieve inversione di tendenza della crescita dell'economia italiana. A questa incertezza di fondo, che caratterizza oggi la situazione economica, il Governo Meloni vuole anteporre una certezza: la certezza di una politica economica sostenibile, che questa NADEF mette nero su bianco in ogni pagina del Documento che stiamo discutendo; la certezza di una politica capace di ridare respiro e slancio all'economia nazionale e di assicurarle perciò un maggiore grado di resilienza. È un'ambizione, visto il periodo che stiamo vivendo, che non dovrebbe trovare divisioni tra centrodestra e centrosinistra, tra maggioranza e opposizione, perché più crescita, più riforme e più investimenti riusciremo a produrre in forma endogena nel nostro Paese e più saremo strutturati per rispondere alla volatilità, all'incertezza e anche al cambiamento dei prezzi relativi che probabilmente ci saranno in futuro. futuro. La crescita diviene variabile fondamentale, via maestra per garantire la sostenibilità del debito, l'equilibrio sociale ed economico e la coesione sociale del nostro Paese. Il ministro Giorgetti lo ha sottolineato ampiamente: questo aggiornamento del Documento di economia e finanza segue un approccio prudente, serio, realistico e sostenibile, vedendo la luce in una situazione economica e di finanza pubblica più delicata di quanto prefigurato la scorsa primavera. Presidente, al contrario di altri, noi riteniamo che la parola prudenza non abbia un'accezione negativa. La prudenza è l'intelligenza del coraggio, perché il coraggio diventa intelligente quando non ha paura di vestirsi con gli abiti della sicurezza, che non deve essere scambiata per codardia. Prudenza vuol dire non far saltare l'economia di questo Paese e i suoi conti pubblici, semplicemente perché

le parole di Marcello Veneziani, che così, dalle colonne di un noto quotidiano, titolava: *spread* significa "scusa per rovesciare Esecutivi antipatici destrorsi". Lo *spread* diviene allora un fantasma che si manifesta solo in presenza di Governi eletti dal popolo, casualmente di centrodestra, ma disprezzati dall'*establishment*, da un certo *establishment*, diciamo. E poi se ne perdono le tracce. Un tempo investì il presidente Berlusconi, facendolo decadere e propiziando l'avvento del Governo tecnico con protettorato a sinistra. Ora accenna a investire il Governo Meloni. Attenzione, però: chi lo dice è complottista e si inventa nemici a scopo preventivo. preventivo. Signor Presidente, al contrario di altri, noi non prestiamo e non presteremo il fianco ai tentativi di destabilizzare l'Esecutivo, frutto della sovranità popolare, che qualcuno magari bolla come un incidente di percorso. Mettere in sicurezza l'Italia e gli italiani è stata la priorità, sin dal primo giorno di Governo; una priorità che si ritrova anche leggendo quegli allegati che, evidentemente, a qualcuno sono sfuggiti. Non è vero, infatti, che l'Italia non spende. La verità è che, sino a questo momento, ha speso male. Lo ripeto: ha speso male. Questo è il coraggio che ha avuto il Governo Governo Meloni: rimettere in ordine i conti per razionalizzare la spesa e passare finalmente a parlare di investimenti. Noi siamo usciti, finalmente, dalla logica dello sperpero e siamo entrati nella logica dell'utilizzo migliore delle risorse economiche della nostra Nazione, come dovrebbe fare un buon padre di famiglia, come si suol dire. Chiedo, allora, a chi quotidianamente critica senza proporre, agitando le paure della gente, dove mai avremmo dovuto metterli i soldi. La verità, onorevoli colleghi, è che in questo momento storico la priorità è il caro energia; la priorità è il carrello della spesa; la priorità è il taglio contributivo; la priorità è adeguare le pensioni al costo della vita; la priorità è tagliare il cuneo fiscale sul lavoro e ridurre la pressione fiscale su famiglie ed imprese; la priorità è accelerare i cantieri PNRR e gli investimenti in infrastrutture strategiche e nazionali; la priorità è gestire e anche contenere i flussi migratori; la priorità è sostenere le famiglie e la genitorialità; la priorità è rinnovare i contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al settore della sanità pubblica, per il quale prevediamo maggiori risorse, non certo tagli come in passato; la priorità è una seria riforma fiscale, una riforma che non strozzi, ma dia invece ampio respiro alle nostre imprese e attragga così maggiori investimenti esteri. La priorità, in estrema sintesi, è evitare il rallentamento dell'economia nazionale. L'Italia deve continuare a poter correre correre veloce. Noi abbiamo un'inflazione che arriva dall'estero. Ciò vuol dire che la nostra economia può tenere, che la nostra economia può reggere e correre. I nuovi obiettivi programmatici contenuti in questa NADEF ci rassicurano. Con la progressiva riduzione dell'indebitamento netto strutturale, il rapporto debito PIL programmatico sarà perciò pari al per cento nel 2023, e così a seguire. Ciò implica che, con lo scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare, si renderanno disponibili spazi finanziari pari a 3,2 miliardi nel 2023, 15,7 miliardi nel 2024 e 4,6 miliardi nel 2025. E nel 2026 il saldo obiettivo sarà riportato al di sotto della soglia del 3 per cento sul PIL. Questa è la serietà che ci chiedono gli italiani. Questo è il pragmatismo di un Governo guidato da Giorgia Meloni. Questa è la credibilità della manovra che ci apprestiamo a varare. Ridurre l'indebitamento netto significherà una sola cosa: dare ossigeno e serenità ai mercati; dare la possibilità di tornare a investire nel Paese, ma soprattutto significherà rimettere in circolo l'economia reale italiana. Mi permetta, signor Presidente, di fare una riflessione e, al tempo stesso, una considerazione politica economica reale. La spina dorsale di questo Paese - come abbiamo visto nei momenti drammatici di crisi economica, come quelli della pandemia - è rappresentata dalle piccole, medie e grandi imprese italiane. La forza del nostro Paese risiede in questo: nell'artigiano, nel libero professionista, nella piccola e media impresa, che si radica sul territorio e che gioca ogni giorno la sfida per la crescita. È la forza di un piccolo eroe comune che ogni mattina si alza, si rimbocca le maniche della camicia e decide di vincere la sfida che la realtà gli pone davanti. Questa è la nostra forza: la produttività, la resilienza e la creatività di questo Paese. È da questo elemento che bisogna partire, con qualsiasi provvedimento di politica economica, per rafforzare e sostenere, in momenti difficili come questo, le nostre imprese, tutte le imprese: quelle piccole, quelle medie, quelle grandi, nonché gli artigiani e i professionisti. Ciò significa non solo investire su di loro, ma anche investire sul futuro del nostro Paese. Così la risorsa pubblica può diventare un moltiplicatore della risorsa privata. Diceva sempre il presidente Berlusconi: senza impresa non c'è ripresa. È ora di lasciarci alle spalle gli interventi economici di stampo assistenzialista che appartengono spesso alla sinistra e inaugurare una nuova stagione, dirottando risorse su quello che non ha funzionato in passato per fronteggiare i rischi di una possibile recessione. Quello delineato dal ministro Giorgetti è perciò un percorso che riteniamo essere virtuoso e che, in modo corretto, tiene conto dell'evoluzione dei saldi della finanza pubblica, con una discesa del *deficit* nominale per effetto delle prossime misure; un percorso che porterà, parallelamente, a un debito pubblico in discesa in rapporto al PIL, nonostante un aumento del debito stesso a fronte del recente ulteriore aumento dei tassi di interesse. Oggi, nel complesso, stiamo cercando di dare un significato importante alla parola "fiducia", che dovrà rappresentare il cuore di un vero e proprio patto per l'Italia. Serve fiducia per aumentare la propensione al consumo e agli investimenti, ma serve fiducia anche per attrarre maggiori investimenti stranieri. Nella manovra economica in via di definizione, una manovra che stimiamo essere di almeno 22 miliardi, la priorità non può essere dunque che accordata a tutte le misure che possono spingere il più possibile sul pedale della crescita. Il Governo ha quindi approntato misure che affrontano i problemi più impellenti del Paese: l'inflazione, la povertà energetica e alimentare, la decrescita demografica, promuovendo al contempo gli investimenti, l'innovazione, la crescita sostenibile e la capacità di reagire dell'economia. avvio a concludere. Quello che viene fatto oggi, con questo atto del Governo che verrà realizzato con la prossima legge di bilancio, è quindi delineare un nuovo approccio, un nuovo metodo di accostamento ai problemi del Paese. Per anni siamo stati costretti a rincorrere le emergenze; da oggi entriamo nella fase di programmazione. In questo primo anno di Governo stiamo gettando le basi non solo per affrontare concretamente i problemi che l'Italia si trascina da anni, ma anche per costruire l'Italia del domani, un'Italia migliore di quella di ieri. Al Governo va il merito di aver tracciato un sentiero sicuro verso questo obiettivo. Signor Presidente, Governo, colleghi, come hanno osservato numerosi analisti, il *vulnus* di questa Nota di aggiornamento sta nelle previsioni di riduzione del debito. È una NADEF che cammina sul filo e in cui, per tener fede ai tendenziali, ogni cosa dovrà andare al suo posto, a partire dalle privatizzazioni, con un'attesa di 20 miliardi entro il 2026: un obiettivo alquanto impegnativo e tutto da verificare. Questo lento calo del debito è già stato recepito dagli investitori, come dimostra non solo lo *spread*, che viaggia stabilmente attorno ai 200 punti base, ma anche i tassi di interesse sui titoli decennali che, per la prima volta dal 2012, hanno toccato i 5 punti percentuali. Ma c'è di più: come è emerso ieri in Commissione, le stime qui contenute sono già superate dagli effetti del conflitto in Medio Oriente, con la necessità di rivedere i saldi di finanza pubblica in una ulteriore ottica prudenziale. A fronte di questa situazione, il Governo sceglie la strada dello scostamento di bilancio, cioè di un ulteriore debito per finanziare circa due terzi della manovra economica. È una decisione, questa, su cui nutriamo diverse perplessità. La prima riguarda la legittimità della richiesta: la Costituzione dice con estrema chiarezza che il ricorso all'indebitamento è consentito solo davanti a una grave recessione economica o a eventi straordinari fuori dal controllo dello Stato. Ma nella Nota di aggiornamento di tutti questi presupposti non vi è traccia; anzi, si sottolinea come anche nello scenario più avverso l'economia italiana sarà comunque in crescita. La seconda perplessità riguarda l'uso che si intende fare delle risorse, ossia la conferma del taglio del cuneo fiscale e la semplificazione delle aliquote Irpef: entrambe le misure sostengono in modo molto limitato la domanda interna e non hanno alcun effetto moltiplicatore sull'andamento economico; sono quindi interventi che non aiutano lo sviluppo e la crescita e che quindi, in prospettiva, non concorrono alla riduzione del debito. Un ulteriore indebitamento, invece, dovrebbe servire per affrontare il drammatico problema del lavoro malpagato o sottopagato, offrendo una risposta concreta ai circa 3 milioni di lavoratori che vivono sotto la soglia di povertà. E dovrebbe servire per proteggere e tutelare la sanità pubblica, che in troppe Regioni sconta il drammatico problema delle liste d'attesa, con un numero sempre maggiore di malati che è costretto a pagarsi le prestazioni. L'aspetto che più ci preoccupa è quello legato al PNRR: mentre in Paesi come la Spagna e il Portogallo sta incidendo positivamente sul PIL, tanto che il Portogallo ha uno *spread* che è la metà del nostro, da noi è praticamente scomparso. La Nota di aggiornamento non dà informazioni sull'andamento della spesa effettiva per l'anno in corso né sull'andamento atteso a partire dal 2024. Allo stesso tempo il Governo continua a parlare di una piena messa a terra delle risorse, ma - cito l'Ufficio parlamentare di bilancio - «In un contesto di inasprimento delle condizioni di accesso al credito, affinché lo stimolo all'attività produttiva sia significativo e duraturo, occorre avanzare speditamente con l'attuazione degli interventi e con le riforme strutturali». In sostanza, se vogliamo che il PNRR sia un fattore di crescita, serve un forte scatto in avanti, non solo sulla capacità di spesa, ma anche sulla messa a terra delle riforme, a cominciare da quelle sulla competitività. In conclusione, Presidente, apprezziamo l'approccio responsabile del ministro Giorgetti e la sua opera di persuasione nei confronti degli altri Ministri, ma allo stesso tempo vediamo un Governo che, a fronte dei rischi fin qui enunciati, non interviene con decisione sull'evasione fiscale e, anzi, manda da più di un anno messaggi di segno opposto, perché se in un anno fai tredici piccoli condoni fiscali, stai dicendo agli evasori che non hanno troppo di cui preoccuparsi. Vediamo un Governo che sul PNRR non solo rallenta attraverso la riforma della *governance* e la rimodulazione della spesa, ma che è ben lontano dal fare le riforme sulla competitività, come ben dimostra la vicenda dei balneari. C'è, in conclusione, molto di cui preoccuparsi e non solo per il contesto generale, ma anche per un indirizzo di questo Governo che non va nella direzione necessaria. Un'ultima precisazione è che normalmente la diligenza del buon padre di famiglia è una diligenza media, ma allo Stato e al Governo è richiesta non la diligenza media, bensì una diligenza molto superiore e molto più incisiva, nell'interesse del Paese.

lo scostamento di bilancio come una strada obbligata, attribuendone la responsabilità alla guerra in Ucraina e alla classificazione dei crediti Eurostat legati al superbonus. - ci dice il Governo - saranno impiegate per confermare il taglio del cuneo fiscale contributivo, continuando così a garantire a lavoratori e lavoratrici gli aumenti attualmente previsti fino a fine anno. Il Ministro ha poi dichiarato che questo si fa soltanto per mettere in busta paga qualcosa, per fronteggiare questo tipo di crisi, ai lavoratori con stipendi più bassi. Lo anticipo subito: il motivo per il quale voteremo contro lo scostamento di bilancio è che non crediamo affatto che lo scostamento di bilancio sia una strada obbligata. Pensiamo che per fronteggiare la crisi che sta pesando in maniera insostenibile proprio sulle fasce di popolazione più fragili, con i redditi più bassi, spesso bassissimi, si sarebbe dovuto intervenire in tutt'altro modo. Lo scostamento di bilancio non sarebbe stato una strada obbligata se si fosse deciso di intervenire in modo deciso, ad esempio sulla questione degli extraprofitti delle grandi imprese del settore energetico, farmaceutico, assicurativo e bancario, quelli che più di altri in questi ultimi anni hanno tratto profitti smisurati di fronte alla crisi. Non sarebbe stata una strada obbligata se si fosse intervenuti per combattere davvero l'evasione fiscale; e parliamo di 100 miliardi, non di spiccioli. Invece, si è deciso di premiare gli evasori, rassicurandoli con condoni e concordati fiscali, diventati ormai sistematici. È un anno che sentiamo questo Governo lamentarsi delle pesanti conseguenze della crisi energetica dovuta al conflitto russo-ucraino, ma non si è fatto nulla di concreto per aumentare l'indipendenza energetica del Paese. Questa secondo noi è una priorità assoluta che si dovrebbe perseguire, avendo le giuste e doverose attenzioni,

Perciò avremmo dovuto e potuto investire su strumenti di fiscalità ambientale. Invece, nonostante tutto, si decide di non investire sulle fonti rinnovabili

per circa 20 miliardi di euro, ben 15 dei quali sono relativi alle fonti fossili, il cui danno ambientale è indiscutibile; fondi che potrebbero essere destinati a interventi di riqualificazione, messa in sicurezza del territorio, rigenerazione urbana delle città. Di tutto questo nell'azione di governo non c'è nulla. La NADEF descrive una situazione di evidente difficoltà, di fronte alla quale questo Governo si sta mostrando del tutto inadeguato, come ha scritto nero su bianco la Corte dei conti nella relazione esposta durante le audizioni dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato, nel corso delle quali ha manifestato tutti i propri timori in merito al quadro che emerge e ai rimedi che paiono timidi e poco efficaci. manifestato preoccupazione davanti alla situazione in cui versa la sanità pubblica: ci sono i problemi legati al reperimento del personale sanitario, alla necessità di bloccare i casi di fuga dal lavoro pubblico;

l'aumento del divario, che evidenzia le differenze tra Regioni; tali differenze non sembrano assorbite, ma al contrario il divario fra alcune Regioni del Mezzogiorno e altre del Settentrione appare sempre più acuto. Garantire i livelli essenziali di assistenza è una priorità cui il Governo sembra indifferente. La condizione in cui versa il Servizio sanitario nazionale imporrebbe un aumento delle risorse pari almeno a 5 miliardi all'anno rispetto a quanto già programmato per i prossimi dieci anni. La situazione è la stessa per quanto riguarda l'istruzione: invece di investire nei giovani, nel futuro di questo Paese, di fronte ai numeri della dispersione scolastica, così così come al disagio giovanile, sembra che questo Governo riesca a intervenire solo con sanzioni, o meglio con sanzioni penali. Il motivo è chiaro: imporre sanzioni è *gratis*, non comporta costi per lo Stato. Molto più dispendioso sarebbe invece investire davvero nella scuola, nella formazione; i soldi impiegati nell'istruzione sono un investimento nel futuro e non possiamo farne a meno; invece, come ho già detto prima, si interviene con delle sanzioni, per di più penali. Ancora, si fa un gran parlare di natalità, della necessità di intervenire per invertire la tendenza all'invecchiamento della popolazione, certificata adesso anche da Eurostat, secondo cui l'Italia è il Paese più anziano in Europa, con un'età media dei suoi cittadini di quarantotto anni. Volete incentivare la natalità, ma poi fate la guerra all'immigrazione, cioè non c'è traccia di una politica di flussi,

questo non è governare, ma vivacchiare sperando che le cose prima o poi vadano per il meglio, aggiustandosi da sole. Questo non succederà, è indispensabile una netta inversione di marcia, del tutto assente nelle intenzioni di Governo. Per questo motivo dichiaro il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

rappresenta lo stato di salute dei conti pubblici, cioè la relazione sul tasso di indebitamento e sul PIL e serve a dirci, in sostanza, come stanno andando le cose, ossia se le previsioni di spesa sono rispettate oppure se qualcosa si sta modificando strada facendo. Volendo mutuare il linguaggio dalla medicina generale - non a caso scelgo questa metafora - potremmo paragonare la NADEF alla cartella clinica del paziente che si sottopone a un *check-up*, all'esito del quale i medici gli diranno se il suo stato di salute è stazionario, se è migliorato o se addirittura è peggiorato peggiorato e nel nostro caso, purtroppo, il paziente Italia è peggiorato. Comprendiamo ovviamente - per sgomberare immediatamente il campo da pregiudizi - che lo scenario internazionale proietta una situazione di grave instabilità economica e finanziaria alla quale si contrappone la necessità per il Governo di far rientrare i conti secondo i parametri dettati dall'Europa. Ma, ciònonostante, riteniamo che questa NADEF sia affetta da due gravi problemi: una rappresentazione ingiustificatamente ottimistica della riduzione del debito negli anni 2024 e 2025, alla quale fa fronte l'affidamento, da parte del Governo, di tutte le risorse per far riprendere la crescita sui fondi del PNNR e, oltretutto, un fantomatico piano di privatizzazione che Bankitalia ha bollato come ambizioso e di dimensioni mai viste prima d'ora. Lo stato delle finanze pubbliche è peggiorato, ma soprattutto quello che non ci piace e che desideriamo mettere in evidenza sono le ragioni per le quali si è verificato questo peggioramento. Certamente ci sono alcuni fattori esogeni. L'aumento del costo delle materie prime e dell'energia, il calo delle esportazioni, l'aumento dei tassi deciso dalla BCE e lo scenario di guerra sono i fattori esogeni richiamati dallo stesso Governo, ma non sono soltanto questi i fattori che determinano questo scostamento. Ci sono dei fattori interni che dipendono dalle scelte che ha compiuto il Governo in questo anno e sono fattori ascrivibili ai provvedimenti che questo Governo ha approvato il più delle volte tramite conversione di decreto-legge e molto spesso ricorrendo alla fiducia, di cui quindi è responsabile. Leggendo la relazione di accompagnamento alla NADEF redatta dall'Ufficio parlamentare di bilancio, emergono due dati sui quali ritengo necessario richiamare l'attenzione. Il primo è la crisi delle famiglie e delle imprese che subiscono l'aumento del costo del ricorso al credito, la perdita del potere di acquisto e l'aumento del costo dei beni primari, come i generi alimentari e dei servizi essenziali, come la sanità (ci arriviamo subito). L'altro dato, invece, riguarda l'occupazione, che resta stabile nel secondo trimestre nonostante la riduzione delle ore lavorate, ma quello che ci dice l'Ufficio parlamentare di bilancio è anche che il costo del lavoro aumenta per unità di misura, quindi

non hanno i soldi, che continuano a perdere risorse e potere di acquisto sul mercato. *(Applausi)*. Come facciamo ad approvare una NADEF, a dire di sì a un Governo che di fronte a questo scenario, che lo stesso Ufficio parlamentare di bilancio ha tracciato in maniera chiara, decide di ridurre la spesa per la sanità di due miliardi, compiendo una riduzione che non è soltanto ingiustificata, ma anche sperequativa, perché chiaramente quelli che non potranno permettersi il ricorso alla sanità privata saranno sempre le stesse famiglie che hanno perso potere di acquisto sul mercato e saranno quelle famiglie che, perdendo la possibilità di rivolgersi alla sanità privata, dovranno attendere nove-dodici mesi per un esame di diagnostica preventiva o che rinunceranno a farlo del tutto. *(Applausi)*. Questo, oltre ad essere un dato umano che non è trascurabile, è anche un dato economico, perché la riduzione delle spese sulla prevenzione prevenzione sanitaria si traduce, nel lungo termine, in un aumento della spesa in termini di costi sanitari per il ricovero, per i contributi di invalidità e di previdenza sociale, oltre che per una progressiva diminuzione anche dell'attesa di vita, perché purtroppo i cittadini che non possono ricorrere alle cure sanitarie sono cittadini che vedono accorciarsi la loro speranza di vita. È anche dispiaciuto veramente assistere all'audizione del ministro Giorgetti, al quale è stato chiesto di indicare come il Governo pensa di far fronte a questa riduzione della spesa e che in sostanza non è riuscito a spiegarcelo. È triste vedere che un Governo non sa come affrontare uno dei problemi più importanti, cioè quello della sanità, così come non ci convince neanche l'aumento delle imposte indirette di circa 14 miliardi a fronte di una riduzione dell'imposizione fiscale diretta di 4 miliardi. Non ci convince perché l'imposizione indiretta è anche questa una misura sperequativa, perché colpisce indiscriminatamente tutte le fasce di reddito ma grava ovviamente di più sulle fasce di reddito basso e medio-basso, cioè sempre su quelle famiglie che hanno perso potere di acquisto, che hanno difficoltà a fare ricorso al credito, che hanno difficoltà a rivolgersi alla sanità e che adesso sono anche gravate da maggiori imposte indirette. Inoltre, non ci convince l'assenza di misure specifiche a favore dell'occupazione, per favorire misure di detassazione e decontribuzione per le imprese che assumono, diciamocelo chiaramente, leggiamo questi dati in maniera integrata - se l'occupazione registra un *trend* positivo, dipende anche dai settori produttivi che in questo ultimo periodo sono riusciti, con l'aumento di risorse, ad assumere. Mi riferisco soprattutto all'edilizia e ovviamente mi riferisco al superbonus, sì, però, rispetto al DEF, il peggioramento del disavanzo del 2023 deriva dalle maggiori spese per i *bonus* edilizi emersi dal monitoraggio in corso d'anno. Detto più semplicemente, senza la spesa per l'erogazione dei contributi del superbonus, la stima del *deficit* sarebbe risultata inferiore a quanto atteso nel DEF, di quattro decimi di punto percentuale di PIL per il venire meno degli interventi del PNRR relativi principalmente agli investimenti. Cioè, lo dico ancora più chiaramente: le risorse del PNRR sono stimate in 200 miliardi da spendere però entro due anni, entro il termine del 30 giugno 2026. Nel 2026 il *deficit* aumenterà oltre che per effetto del effetto del trascinamento delle imposte dirette, anche per la ritardata realizzazione di interventi del PNRR *(Applausi)* cui si aggiungono gli effetti, divenuti sfavorevoli, dei *bonus* edilizi. Allora è evidente che questa NADEF fotografa una situazione di assoluto allarme, dove i *bonus* edilizi aumentano la spesa e l'indebitamento da un lato e le previsioni di contenimento del *deficit* derivano soltanto dalle risorse del PNRR che però, attenzione, dobbiamo spendere entro il 2026, altrimenti dovranno essere restituite restituite e si tradurranno in un ulteriore debito per l'Italia. Questa, Presidente, non è la nostra opinione, ma è quanto ha evidenziato la stessa Banca d'Italia che ha formulato un chiaro avviso al Governo, richiamando la sua attenzione sul fatto che quanto più la crescita beneficia delle misure contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, tanto più è necessario il massimo impegno per la sua tempestiva attuazione, salvaguardando gli obiettivi complessivi ed evitando di accumulare ritardi. In conclusione, questa NADEF fotografa un *deficit* che sale al 5,3 per cento nel 2023 per effetto della contabilizzazione del superbonus e che sarà fissato nel quadro programmatico al 4,3 nel 2024. Il Governo, dunque, prevede di peggiorare il disavanzo sia per l'anno in corso che ulteriormente per l'anno successivo e una ulteriore riduzione la prevede per gli anni successivi. Dunque, questa NADEF 2023 non ci convince, perché le soluzioni che propone al fine di contenere il *deficit* pubblico non ci appaiono risolutive e soprattutto non comprendiamo, perché non è indicato, dove verranno trovate le risorse e come e quando verranno impiegate. Il Governo ci dice che intende adottare determinate misure che rinvia alla legge di bilancio, l'adozione di misure per la riduzione del cuneo fiscale, per l'attuazione della prima fase della riforma fiscale, per introdurre misure di sostegno alle famiglie, per la prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, per il potenziamento degli investimenti pubblici e per il finanziamento di altre misure già previste negli anni precedenti. Tutto bello a parole, tutto molto convincente, tutto sicuramente entusiasmante, ma sono misure che non ci convincono e sulla cui attuazione lo stesso Governo non sa come fare, perché l'unica risorsa economica immediatamente disponibile, come ho già detto, dipende dai fondi del PNRR, che questo Governo ha già rimodulato e di cui quindi si deve assumere pienamente la responsabilità dell'attuazione e che invece, come la stessa Banca d'Italia ha evidenziato, rischia di rimanere inattuato, generando nuovo debito, insostenibile debito. Non ci convince neanche il programma di privatizzazioni di cui non viene fornita neanche una descrizione. Non si capisce che cosa riguardino, ma è sempre Bankitalia a bollarlo come il piano più ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato. Ci sembra che sia già di per sé allarmante e poco credibile. Non ci convince, infine, perché questo Governo continua a favorire misure per l'occupazione temporanea e non incide sulla detassazione dei posti di lavoro, che sarebbe l'unica misura per consentire alle imprese di assumere e far ripartire la crescita. In conclusione, Presidente, riprendendo la metafora iniziale, il paziente Italia sta peggiorando e la cura proposta dal Governo non è in grado di salvarlo. Per queste ragioni, Presidente, il Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope esprime un voto contrario sulla

dello scorso anno sulla base di numeri e scelte in gran parte ereditati dal Governo precedente, ma soprattutto frutto di inevitabili compromessi tra forze politiche molto diverse tra loro. Quella manovra, seria e responsabile, venne approvata da tutti, lodata dall'Europa, avviando un lavoro preciso e puntuale di revisione del PNRR per rimediare alle lacune ereditate. Per inciso, chi oggi continua a raccontare agli italiani bugie dei tagli del PNRR e delle risorse perse, dovrebbe scusarsi e congratularsi con il Governo per l'ennesimo traguardo raggiunto poche ore fa con l'erogazione della terza rata, che rappresenta una vittoria per tutta l'Italia. Per fare chiarezza ricordo che i giorni della manovra hanno visto un periodo difficile con i costi dell'energia ai massimi storici, le famiglie e le imprese in sofferenza per l'inflazione in continua crescita. Ricordo il Governo impegnato a concludere nel più breve tempo possibile in sede europea l'accordo per il tetto al prezzo del gas. poi seguiti mesi di scelte coraggiose; ricordo tra tutte l'abolizione del reddito di cittadinanza, l'introduzione di una netta e sacrosanta distinzione tra chi non è nelle condizioni di lavorare e, quindi, deve continuare continuare a ricevere dallo Stato un aiuto concreto e chi, invece, a lavorare ci può andare. *(Applausi)*. Sono stati mesi di dati *record* sul fronte dell'occupazione che ha raggiunto numeri straordinari e, contrariamente alla falsa narrazione della sinistra, sulla precarizzazione dei rapporti di lavoro ha visto la crescita di contratti stabili e dell'occupazione giovanile. Sono stati mesi in cui il Governo e la maggioranza hanno varato quella rivoluzione fiscale che prenderà corpo prima della fine del mandato; una riforma strutturale che taglia le tasse a famiglie e imprese e ricostruisce il rapporto tra cittadino e fisco all'insegna della fiducia e non del sospetto. Una grande battaglia storica di Forza Italia, il grande sogno liberale del presidente Berlusconi *(Applausi)*, che noi vogliamo portare a compimento entro il termine di questa legislatura. Sono stati però anche mesi nei quali le condizioni esterne non sono migliorate; la BCE ha continuato a somministrare al paziente europeo affetto da alta inflazione la medicina sbagliata, continuando ad aumentare quei tassi di interesse che stanno strozzando le famiglie, frenando gli investimenti delle aziende e creando un effetto potenzialmente recessivo. La locomotiva tedesca si è fermata; la Germania è di fatto in recessione tecnica, trascinando inevitabilmente verso il basso le altre economie europee a partire da quelle più interconnesse proprio come la nostra. La guerra in Ucraina continua a palesare i suoi effetti devastanti e anche a causa delle vicende recenti del fronte mediorientale, con la brutale aggressione di Hamas contro Israele, la situazione economica internazionale potrebbe ulteriormente complicarsi. Nel frattempo si è manifestato in tutta la sua drammaticità il peso delle scelte fallimentari, per non dire disastrose del Governo giallorosso, che ha aumentato a dismisura il debito pubblico, terremotando le finanze pubbliche. Ecco dunque come arriviamo a questa NADEF e alla legge di bilancio che il Governo si appresta a presentare la prossima settimana. Il quadro di finanza pubblica che la NADEF delinea riflette ancora una volta un'impostazione prudente, con una leggera revisione delle stime di crescita per il 2023-2024, a causa del rallentamento dell'economia che stiamo vivendo. è proprio questo rallentamento, insieme all'andamento dell'inflazione, a richiedere di continuare con una politica di sostegno ai redditi e alle pensioni più basse. Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo contributivo sul lavoro e sulle pensioni e all'attuazione della prima fase della riforma fiscale, la pressione fiscale nel 2024 inizierà il suo percorso di riduzione. Le tasse scenderanno e verranno rafforzati gli interventi a favore delle famiglie e della natalità, perché fare figli non deve essere più considerato un lusso o un'incoscienza, ma il più grande investimento sul futuro della Nazione. Si interverrà sul rinnovo dei contratti pubblici ancora bloccati, a partire dal comparto sanità, che in questi giorni è stato utilizzato come clava dall'opposizione contro il Governo, usando la salute per cercare di fomentare il malessere sociale. Riuscite a dare la colpa a questo Governo se per fare una mammografia ci vogliono sei-otto mesi, dimenticando di raccontare che non avete fatto programmazione sanitaria in questi dieci anni in cui avete governato come azionisti di maggioranza, lasciandoci un'eredità e un fondo sanitario insufficiente e un'organizzazione inefficiente e obsoleta. *(Applausi)*. E poi - permettetemi - si è superato il ridicolo. Prima ancora di sapere quanti soldi il Governo stanzierà in legge di bilancio per la sanità, la sinistra ha cominciato a gridare ai tagli e all'assalto della destra alla sanità pubblica. Peccato che i numeri dicano tutt'altro e chiariscano in maniera inequivocabile che nei prossimi anni i fondi per la sanità non diminuiranno, ma aumenteranno, per dare *in primis* una risposta al problema che sta più a cuore agli italiani: le liste d'attesa. La maggioranza sta già lavorando ad una vera riforma sanitaria. Quello che invece verrà sicuramente tagliato saranno gli sprechi e i privilegi: non un solo euro dei cittadini italiani verrà sprecato in politiche assistenziali. Si tornerà a parlare di privatizzazioni e di valorizzazione degli *asset* pubblici sottostimati, come noi di Forza Italia chiediamo con forza, per andare a ridurre lo *stock* del debito e aumentare la fiducia degli investitori nella volontà politica del Governo e della maggioranza di proseguire nel percorso di contenimento di *deficit* Le ironie che ho ascoltato sui 23,5 miliardi di scostamento di bilancio che ci apprestiamo a votare sono decisamente fuori luogo, soprattutto da parte di chi - come ho già detto - ha sulla coscienza la responsabilità di quel buco che oggi ci obbliga a investire in *deficit*, un *deficit* indispensabile. Chi ci critica dovrebbe riconoscere che l'alternativa allo scostamento sarebbe stata una manovra lacrime e sangue, cioè una manovra di tagli che, unita alla politica monetaria restrittiva della BCE, avrebbe significato incidere sulla carne viva degli italiani. Dico di più: questo lavoro serio e responsabile ci consente oggi di sederci a Bruxelles, per la trattativa sulla riforma del Patto di stabilità e crescita, con le carte in regola. E voglio chiudere su questo: sostenere il Governo in questo negoziato dovrebbe essere il minimo sindacale per ogni forza di opposizione che abbia a cuore il futuro dell'Italia. Noi di Forza Italia siamo convinti che l'Unione europea debba essere coerente con gli investimenti che chiede ai suoi Stati membri. Non Non ha alcun senso che investimenti come quelli sulla transizione verde e digitale o sulla difesa vadano ad accumularsi al nostro debito, che è già ingente. Sarà una battaglia difficile, con schieramenti trasversali alle diverse famiglie politiche europee; avremo bisogno della massima coesione nazionale possibile. Ci auguriamo che la sinistra rifletta su questo e intanto noi continuiamo a lavorare, applicando le tre "T": talento, tolleranza, tenacia. Questo Governo ha talento, dimostrato dalla capacità di vedere oltre la crisi, tolleranza, verso chi lo attaccava con pregiudizi e ancora oggi verso chi racconta al Paese una realtà diffamatoria, e tenacia, la tenacia di chi lavora sodo per dimostrare con i fatti capacità e competenza, la tenacia di chi sa che non sarà facile, perché ha davanti a sé una montagna da scalare, guardando avanti e puntando con decisione e sicurezza alla vetta. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

una questione. Non credo che il Presidente del Consiglio debba per forza seguire i lavori di quest'Aula in tutte le sue manifestazioni. Non credo che il Governo debba essere schierato al completo ogni volta che si tratta un qualsiasi argomento. È, però, inaccettabile che, a parte il ministro Ciriani, che è appena entrato in Aula, non ci sia un solo Ministro della Repubblica italiana quando si discute della NADEF e che il ministro Giorgetti non abbia messo piede in quest'Aula fino a questo momento. *(Applausi)*. Ciò dimostra una cultura delle istituzioni che, evidentemente, questo Governo non ha. Non solo non c'è la presenza: in Commissione bilancio il Governo non ha replicato agli interventi dei colleghi in quest'Aula, il relatore e il Governo non hanno replicato sul documento, uno dei più importanti, che prelude alla legge di bilancio e che riguarda il Paese nella sua interezza. Anche questo, a mio parere, è assolutamente inaccettabile. non c'è molto da dire. Siamo, a mio avviso, di fronte ad un vero miracolo, perché ci vogliono doti sovrumane per un Governo che era pronto, che ha ereditato un biennio di crescita al 12 per cento e che riconsegna, dopo un solo anno di lavoro, un valore del più 0,8, con una previsione del tutto ottimistica, perché molto probabilmente questo dato sarà più negativo di quanto ho appena detto.

il rapporto debito-PIL, nonostante quello che si è detto in questi giorni, nell'ultimo triennio, cioè dal 2021 ad oggi, a fine 2023, cala di quindici Il rapporto debito-PIL è calato di quindici punti. Voi, invece, riconsegnate un Paese in cui il debito in rapporto al PIL non calerà nei prossimi anni.

Perché i dati macroeconomici si valutano in frazione: il rapporto *deficit*-PIL ed il rapporto debito-PIL. Ed è evidente che una spesa non può essere valutata soltanto come dato oggettivo, ma in funzione della crescita che comporta. però, su questo più avanti. Abbiamo lasciato anche il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Io non penso che siano stati tagliati i fondi dalla Commissione, che non ha erogato cifre nella terza rata. No, le risorse le ha tagliate questo Governo, nella revisione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, che taglia sedici miliardi rispetto al dissesto idrogeologico, alle periferie e alle spese dei Comuni, che tra l'altro amministrate molto spesso voi e che ritenete non siano in grado di completare Governo ha ereditato una situazione molto favorevole. E non possiamo certo dire che non ci fossero problemi prima di questo Governo, perché noi abbiamo affrontato una pandemia e l'inizio della guerra in Ucraina. La colpa, ovviamente, è sempre di qualcun altro. Come dicevo, nel triennio successivo alla pandemia, il rapporto debito-PIL è sceso di media di cinque punti percentuali l'anno. Ora, se tutto va bene, scenderà in media dello 0,2 all'anno: cioè il 96 per cento in meno. È un Governo che ha ereditato, come certificato peraltro dall'ultimo Rendiconto generale dello Stato approvato da quest'Aula, un Paese che ha segnato 100 miliardi di euro di gettito fiscale in più, frutto, anche e soprattutto, del superbonus che ha fatto emergere ogni euro di evasione fiscale nel settore dell'edilizia. Peraltro, sul tema del superbonus io ricordo, per onestà intellettuale, ciò che ha dichiarato poche ore fa il ministro Giorgetti: io ero qui anche quando il debito si è avvicinato per un pelo al 100 per cento del PIL. Cosa è successo non è colpa né di Berlusconi né di Conte. C'è stato il caso Lehman Brothers e c'è stato il Covid-19. È in quelle circostanze che il debito schizza e prende venti punti di PIL ogni volta. Questa è la verità. Togliete l'effetto *shock* dei due fattori esogeni, che non dipendono dal controllo della politica italiana, e avrete, probabilmente, un profilo di debito diverso rispetto a quello che abbiamo oggi. Non posso che ringraziare il ministro Giorgetti, peraltro uno dei pochi che si è sempre schierato contro il superbonus e che non ha cambiato idea. Vedo tantissimi membri di questa maggioranza, che nello scorso Governo chiedevano proroghe, che in questo Governo si fanno approvare ordini del giorno per richiedere la proroga del superbonus e poi dicono che è la più grande truffa dello Stato. *(Applausi)*. Ci sono altri passaggi meravigliosi che voglio segnalare, li leggo: leggo: la legge Fornero, elevando i requisiti di accesso per il prepensionamento, ha migliorato in modo significativo la sostenibilità del sistema pensionistico nel medio e lungo periodo, garantendo una maggiore equità tra le generazioni. È un elogio alla legge Fornero scritto nella NADEF che stiamo votando; non mi sembra che la Lega abbia mai avuto questo tipo di posizione sulla legge Fornero, ma questa è la posizione del ministro Giorgetti. È una NADEF che, dopo essersi arresa al crollo della crescita del 2023, spara una previsione comunque non lusinghiera di un +1,2 per cento del 2024, a dir poco ottimistica, visto che le ultime previsioni del Fondo monetario internazionale, dell'OCSE, della Commissione UE e di Prometeia oscillano al massimo tra un +0,4 per cento e un +0,8 per cento. Insomma, previsioni a casaccio, nessuna visione di politica industriale, nessuna soluzione ai tanti problemi che attanagliano famiglie e imprese di questo Paese. Avete tolto il motore economico del Paese, eliminando il superbonus e transizione 4.0, e l'avete sostituito con "Gli appunti di Giorgia", che mi sembra siano carta straccia. Quando ho sentito dire - è accaduto molto spesso - da questa maggioranza e in particolare dal Presidente del Consiglio di lasciare in pace chi vuol fare, rivolgendosi agli imprenditori, avevo la preoccupazione che si lasciasse fare veramente un po' tutto, ma la speranza era che in qualche modo ciò si accompagnasse a una ripresa economica sostenendo le esigenze dell'impresa.

Per quanto riguarda l'espansività della legge di bilancio (che è stata spacciata come espansiva perché ci sono 15 miliardi in *deficit*), credo che non ci si possa nascondere dietro il fatto che che uno scostamento di bilancio c'è, dal punto di vista delle opposizioni, perché è del tutto inadeguato rispetto alle esigenze del Paese. Annuncio quindi che anche sulla Relazione al Parlamento il MoVimento 5 Stelle voterà contro, perché lo riteniamo insufficiente e perché pensiamo che non vada a toccare i punti necessari di sostegno al nostro Paese.

e che non dà un euro in più rispetto a quanto previsto nel 2023, già totalmente eroso dall'inflazione che sta dilagando nel nostro Paese. Certo, è colpa della BCE, ma poi qualcuno magari ci dirà chi ha il controllo della BCE, chi ha quote importanti della BCE, chi parla con la BCE. La Banca La credibilità di questo Governo si misura anche sulla capacità di andare in Europa con gli interlocutori europei e ottenere qualcosa per questo Paese, cosa che non sta succedendo su nessun fronte.

quando si parla di superbonus, si guarda soltanto la spesa e non il rapporto debito-PIL e *deficit*-PIL creato dal superbonus; quando invece si parla di spesa sanitaria, si guarda soltanto in rapporto al PIL e alla crescita storica. Non ho ben capito perché si usano due pesi e due misure prima delle quali è il tema delle privatizzazioni: sono davvero basito, perché è surreale che in questo Paese si parli di privatizzare Ferrovie

totale austerità. I principi dell'austerità, che sono pochi, sono le privatizzazioni, l'avanzo primario e la precarizzazione del lavoro. I dati sul numero di occupati sono molto buoni, certo, ma qual è la qualità di quel lavoro, grazie alle vostre politiche? Insomma, Presidente, questa NADEF è un disastro e noi ovviamente voteremo convintamente contro. L'Italia nel frattempo è in stagnazione, ma state tranquilli, perché è tutta colpa del superbonus, è tutta colpa dei benzinai, è tutta colpa della BCE, è tutta colpa dell'Europa e un pochino pure della Wagner.

senatori, parlare di NADEF, così come di DEF, è un rito che non rappresenta, secondo me, uno dei momenti più alti del dibattito parlamentare, perché, come tutti sappiamo, si tratta di documenti inemendabili.

Si potrebbe pensare magari in futuro a cambiare questa prassi, magari a fare in modo che sia data al Parlamento l'opportunità di fare osservazioni al Governo, in modo tale che possa eventualmente recepirle. Al momento però le cose stanno così, per cui non è che ci sia molto da dire. In compenso, però c'è molto da leggere. Qual è la cosa che a me piace molto invece della NADEF e del DEF? È che si parla di numeri e i numeri quelli sono e rimangono a futura memoria: quindi, possiamo tranquillamente andare indietro nel tempo e vedere cosa prevedevano altri Governi e altri Ministri e vedere che cosa poi è successo, perché alla fine - come ho sentito un collega argomentare prima - la NADEF dice lo stato delle cose. Ebbene, questo è lo stato delle cose dopo un anno abbondante di Governo del centrodestra: vediamo se ha fatto meglio o peggio rispetto a quello che altri (quindi non sospettabili di essere di parte) dicevano che sarebbe stato, con numeri in passato validati tra gli applausi dall'Unione europea. Ahimè, cominciamo con l'ultima NADEF fatta dalla strana coppia Gualtieri-Conte. Lo so, amici del Partito Democratico, a me dispiace, ma avete avuto una volta la possibilità di mettere un ministro dell'economia politico

Cos'era il debito pubblico previsto da Gualtieri e Conte per il 2023, validato fra gli applausi dell'Unione europea? Il debito pubblico pubblico tendenziale e programmatico previsto per la fine di quest'anno era il 154 e il 151,5 sul PIL; peccato che noi adesso abbiamo il 142, dopo lo scostamento. Se non facessimo lo scostamento, sarebbe al 140. Stiamo parlando di quasi 15 punti di

Attenzione, perché i numeri sono importanti. Lo stesso PIL era previsto,

Il Ministro dell'economia e il Ragioniere generale dello Stato mica possono sbagliare, quindi i loro numeri saranno sicuramente legge, vangelo: di qui non si sbaglia.

Altrimenti, non mi spiego come, pur in presenza di guerre, la disoccupazione è più bassa rispetto a quello che il migliore prevedeva per la fine di quest'anno.

perché dovremmo dire che in ogni caso i nostri conti sono migliori di qualsiasi aspettativa che era stata fatta anche da quelli bravi. Attenzione, perché il passaggio successivo, vale a dire la validazione da parte dell'Unione europea,

però, guarda caso, quella non andava bene all'Unione europea. Stiamo molto attenti quindi a vedere quale sarà adesso il comportamento dell'Unione europea, perché, se per caso dovessimo scoprire che non contano i numeri, né quello che si fa, ma conta se gli mandiamo un amichetto loro, anche se incompetente come Gualtieri, perché allora approvano tutto,

di elezioni europee diano una bella lezione a questi maestrini che non la prendono mai giusta. *(Applausi)*. Abbiamo un'ottima occasione in sede elettorale per dire come la pensiamo. Nello specifico, giusto per capire cosa potrebbero mai argomentare queste persone che, come alcune volte dico, hanno la scadenza come lo yogurt,

se una frase ha senso, bisogna provare l'opposto. È mai possibile che raccomandino di avere una politica di bilancio imprudente per una crescita insostenibile? Non credo, quindi significa che non ci hanno detto nulla. Direi quindi che abbiamo tutti i numeri per presentarci non a testa alta, ma altissima, con questa NADEF davanti all'Europa, sfidando tutte le persone che vorranno dirci che le cose non vanno bene perché magari qua c'è qualcuno che politicamente non è della loro casa e possiamo tranquillamente portare a casa i risultati di un anno di lavoro nell'interesse degli italiani e che proseguirà ancora in questa direzione.

*(Applausi)*, per mesi di parole ne hanno dette tante e ci hanno raccontato che l'economia italiana andava bene, che facevamo meglio del resto d'Europa e poi a Cernobbio il ministro Giorgetti, che saluto e ringrazio per la sua presenza, ha suonato il contrordine e ci ha detto che l'economia si era fermata e che la coperta era corta. Ora, signor Ministro, non bisognava essere laureati ad Harvard per capire già da tempo che l'inflazione avrebbe ridotto i consumi e che i tassi di interesse e l'incertezza geopolitica avrebbero pesato. Il problema, signor Presidente, è che il Governo ci ha messo del suo, la coperta se l'è un po' accorciata da solo. Bisognava andare avanti sulla lotta all'evasione fiscale e avete fatto quattordici condoni. *(Applausi)*.Serviva fare per tempo la revisione della spesa e avete fatto cassa sui pensionati e cassa sui poveri, eliminando il reddito di cittadinanza e deindicizzando le pensioni. Avete denunciato i costi del superbonus. Certo, è costato tantissimo, molto di più delle previsioni e andava ridimensionato prima,

che il Parlamento ha via via approvato. Grida allo scandalo lo stesso Governo che a febbraio ha bloccato la cessione dei crediti, ci ha raccontato che era tutto sotto controllo e sette mesi dopo si è svegliato dicendo che c'erano 20 miliardi di costi in più. Si è accorciato la coperta, il Governo, con le sue incertezze sul superbonus, con il cambio di *governance*, con la revisione presentata all'ultimo, con i 16 miliardi di progetti definanziati, lasciando in mezzo al guado le amministrazioni locali su progetti che erano in dirittura d'arrivo.

Questi 20 miliardi sono decisivi per la sia pur lieve riduzione del debito fino al 2026. È il triplo di quanto è stato fatto nell'ultimo decennio e ci chiediamo da dove verranno tutti questi soldi, perché per il momento - mi rivolgo al ministro Giorgetti - le scelte del Governo sono quantomeno contraddittorie. Avete deciso di cedere ITA a Lufthansa? Amen, ma sulla rete TIM state mettendo 2,5 miliardi di euro, ma avallando la cessione di un'infrastruttura strategica al 65 per cento al fondo americano KKR. Sull'ILVA dovevate entrare in maggioranza, ma avete cambiato idea e quell'azienda di primaria importanza è nell'incertezza più totale. *Dulcis in fundo*, Ministro, Poste Italiane

perché ci vuole un disegno di politica industriale dietro queste scelte; vogliamo anche capire che idea ha il Governo del ruolo dello Stato, perché, se il tema è fare cassa a prescindere dalla politica industriale, stiamo portando il Paese in una direzione sbagliata. Terzo elemento di fragilità di questa NADEF sono i fattori di rischio, che non sono, purtroppo, improbabili. Riguardo gli interessi sul debito pubblico, andiamo da 78 miliardi a 104 e basta un ulteriore aumento dei tassi per sballare i conti. Pensiamo alle tensioni geopolitiche, pensiamo al PNRR. Il DEF stimava che due terzi della crescita del triennio 2024-2026 sarebbero derivati dall'attuazione del Piano. Sul Piano siamo in ritardo, siete in ritardo e, se la situazione non viene sbloccata, la crescita modesta prevista dal DEF nel 2024-2026 va a farsi benedire. Sono questi i fattori, non un complotto della finanza internazionale, che spiegano il nervosismo dei mercati e lo *spread* che purtroppo è tornato ad avvicinarsi a quota 200. Ora, il cuore di questa manovra è la richiesta di scostamento su cui dovremo votare. È molto rilevante soprattutto per il 2024 e vale circa due terzi della manovra. Sono quattro volte di più di quello che avevate previsto nel DEF. Ora, alcuni colleghi hanno denunciato l'incostituzionalità di questa richiesta di scostamento. Vedremo, direte quello che ne pensate, ma il punto di fondo è un altro, Presidente: il Governo chiede al Parlamento uno scostamento per fare cosa? La cosa più importante è il taglio del cuneo fiscale. Lo condividiamo...

il taglio del cuneo fiscale: è una scelta che condividiamo. Peccato che utilizziate il *deficit* per farlo per un solo anno e senza una copertura certa. Anzi, state di fatto introducendo una nuova clausola di salvaguardia. Il Ministro ha usato il termine ipoteca per i futuri Governi. Secondo, per quanto riguarda la spesa sanitaria pubblica, il tendenziale scende dal 6,6 per cento del PIL al 6,2. Per riportare la spesa a livello del 2023, il vostro livello, servirebbero 7 miliardi in più. Non c'è traccia di questo impegno, se non il tema del rinnovo del contratto di lavoro, che è importante, ma non basta a risolvere i problemi del sistema sanitario pubblico. In terzo luogo, chiedete *deficit* per finanziare la riforma fiscale, ed è una riforma che noi consideriamo iniqua e inadeguata. Non l'abbiamo votata e l'abbiamo contrastata in Parlamento. Voi volete accorpare i primi due scaglioni, cosa che non cambierà di una virgola la situazione di 18 milioni di contribuenti con redditi fino a 15.000 euro *(Applausi),* che sono quelli che avrebbero più bisogno di aiuto, e distribuite a pioggia 3 o 4 miliardi di euro sui 24 milioni di contribuenti rimanenti. Mi avvio alla conclusione, signor Presidente: il ministro Giorgetti ha definito questa NADEF prudente e realista. La verità è un'altra. La verità è che il Governo ha costruito una NADEF fragile e debole; fragile per i motivi che ricordavo in precedenza, perché i numeri sono scritti sulla sabbia, e debole perché inadeguata, non affronta i nodi dello sviluppo e dell'equità sociale. L'Italia avrebbe bisogno di ben altro, di una nuova politica dei redditi, non solo del taglio del cuneo fiscale, una legge sul salario minimo, di una legge sulla partecipazione dei lavoratori e dell'impegno per il rinnovo dei contratti, insomma, misure vere contro il carovita, non il trimestre del ministro Urso. Abbiamo bisogno di rispondere alle istanze del Paese, che si è visto impoverire in questi anni di inflazione. Presidente, il 7 ottobre sono scese in piazza a Roma 200.000 persone. *(Applausi)*. Il Partito Democratico e le altre forze di opposizione hanno raccolto centinaia di migliaia di firme per una legge sul salario minimo. Sono istanze che meritano rispetto e ascolto da parte del Governo, così come merita rispetto e ascolto chi chiede di rifinanziare la sanità e i servizi pubblici essenziali, come la scuola, la ricerca, il trasporto pubblico; ugualmente, merita un'attenzione massima da parte di tutto il Paese l'attuazione degli investimenti e delle riforme del piano. Come ha ricordato anche ieri il presidente Mattarella, Mattarella, il PNRR è un'occasione storica per l'Italia e lo è anche per l'Europa; la sua piena riuscita è un interesse comune, che merita tutto l'impegno e la solidarietà di cui la nostra società è capace. Signora Presidente, la prossima legge di bilancio sarà un banco di prova importante per il Governo e per il Paese. Per un anno ci avete raccontato una realtà immaginaria e avete fatto molta propaganda, ma avete fatto molto poco di quello che era necessario per il Paese. Ora siete costretti a fare i conti con la realtà e la realtà purtroppo è che l'Italia si è fermata e non avete la più pallida idea di come farla ripartire. La realtà è che invece di raccontare e discutere con noi quello che volete fare per il Paese, continuate a fare, senatore Borghi, l'opposizione all'opposizione *(Applausi),* perché è l'unica cosa che sapete dire nelle Aule del Parlamento. Sono questi i motivi per cui il Gruppo Partito Democratico voterà contro lo scostamento e contro la Nota di aggiornamento.

la prassi richiederebbe una dichiarazione di voto argomentata e articolata rispetto alle posizioni del Gruppo Fratelli d'Italia per quanto riguarda questa Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Mi Mi consentirà però, Presidente, qualche riflessione. Ho ascoltato attentamente gli interventi in Aula, in particolar modo quelli della minoranza, in Commissione e anche in audizione. Ringrazio il ministro Giorgetti per l'attenzione ed anche per la pazienza che ha avuto rispetto a esternazioni offensive che ci sono state

geopolitico e una contingenza economico-finanziaria evidentemente nuova per voi. Non vi siete resi conto che c'è ancora una guerra in Ucraina e ci sono ancora conseguenze economico-finanziarie che richiedono lo scostamento di bilancio. Ho ascoltato anche autorevoli esponenti della minoranza chiedere l'incostituzionalità dello scostamento di bilancio, perché ne mancano le condizioni. Non ci sono le condizioni oggi con una guerra ancora in corso in Ucraina, con le conseguenze che ancora paghiamo e con un'ulteriore problematica e un ulteriore conflitto in Israele. Ieri sera eravamo tutti quanti all'Arco di Tito ad esprimere solidarietà al popolo israeliano. Ebbene, benvenuti sulla Terra.

qualcosa che non va e c'è molto spesso un qualcosa di negativo per chi subisce queste decisioni. In un documento economico-finanziario non ci può essere la parola "gratuità", che invece è comparsa nei vostri testi, testi, quando avete convinto l'Italia che si potesse ricostruire l'intero patrimonio edilizio in maniera gratuita. Ebbene, ci sono 80 miliardi da restituire in quattro anni, un debito da onorare, senza il quale il nostro *deficit* sarebbe sceso di un punto l'anno. E questo non lo dice Giorgia Meloni, non lo dice Giorgetti, non lo dice Fratelli d'Italia e non lo dice il senatore Liris. Per voi che siete innamorati dei colossi bancari internazionali, per voi che giocate con frenesia al gioco "forza *spread*", che vi vede sempre protagonisti e citare i colossi economico-finanziari internazionali, ebbene quest'affermazione, queste citazioni, queste puntualizzazioni sono parte di un *report* dettagliato di Goldman Sachs, che il 27 settembre l'ha messo giù in maniera molto attenta e molto ben confezionata, all'interno del quale c'è scritto che l'aumento del *deficit* fiscale è quasi interamente dovuto ai crediti d'imposta sui *bonus* edilizi. Se a questo sommiamo i tassi di interesse della BCE, che hanno bruciato ulteriori 15 miliardi, si compone il quadro della tempesta perfetta, che che oggi constatiamo e sul quale ci misuriamo, su queste difficoltà, su questa contingenza e su questa congiuntura economico-finanziaria e geopolitica,

con gli elettori e con i nostri concittadini, cioè il taglio del cuneo fiscale per tutto il 2024, la riforma fiscale, il sostegno alle famiglie e alla genitorialità,

a parlare per suggestioni e per speculazioni, ma i fatti sono numeri e i numeri sono fatti. E questi sono i numeri di questo Governo, così come è un fatto concreto il rinnovo del contratto nazionale per 135.000 dirigenti medici e non, per quanto riguarda il Servizio sanitario nazionale. altro tassello che il Servizio sanitario nazionale aspettava da tempo. Questa è la dedizione che riserviamo

emendamento per eliminare la follia dei gettonisti, che umiliano il Servizio sanitario pubblico e assorbono tante risorse delle Regioni e dello Stato.

delle affermazioni e dei principi da sostenere con forza. Lo ha detto in audizione: la prudenza è un concetto economico, il realismo è un concetto politico. siamo per questo combinato disposto, che possa essere la soluzione. Ed esso non poteva che suscitarmi un aforisma, una citazione, che più più o meno recita nel modo seguente: il pessimista si lamenta del vento. L'ottimista aspetta che il vento cambi. Il realista aggiusta le vele. Noi siamo quello *skipper* che guarda il mare

la Commissione bilancio, il relatore, presidente Calandrini, e tutti coloro che hanno, con forza e professionalità, portato avanti un'azione di credibilità

facendoli precedere da un minuto di silenzio in ricordo delle vittime di quella

Signor Presidente, sono passati sessant'anni da quella terribile sera del 1963 ed è impossibile dimenticare quel che accadde alle ore 22,43 del 9 ottobre. Dal monte Toc, dietro la diga del Vajont, diga a doppia curvatura, la più alta del mondo, si staccano tutti insieme 260 milioni di metri cubi di roccia che cadono nel lago artificiale e sollevano un'onda gigantesca che, precipitando a valle, spazza via il paese di Longarone e devasta Castellavazzo, Erto e Casso, facendo quasi 2.000 vittime (1.910 dicono le cifre ufficiali). «Scrivo da un paese che non esiste più»: così inizia il *reportage* uscito due giorni dopo su «La Stampa»; a firmarlo è quello che allora era un giovane inviato, Giampaolo Pansa, che già a caldo parla di una tragedia di proporzioni enormi. Un disastro gigantesco sì, ma - come ha voluto ricordare il presidente Mattarella in quei luoghi lunedì scorso - non è stata una fatalità; piuttosto una drammatica conseguenza di precise colpe umane, della devastazione di un territorio stravolto nel suo assetto naturale e sociale. Una giornalista tenace e coraggiosa come Tina Merlin dalle pagine de «l'Unità» aveva denunciato i pericoli che si nascondevano dietro il faraonico progetto della ditta SADE. Ma lo Stato abdicò alle funzioni di controllo e di salvaguardia del territorio e delle popolazioni; gli interessi industriali e finanziari pesarono più di ogni altra considerazione, più delle stesse inchieste. Solo dieci anni fa, in occasione del cinquantesimo anniversario, le più alte cariche delle nostre istituzioni si sono inchinate e scusate per quel che accadde, per le omissioni, per i silenzi e per le responsabilità. Concludo, signor Presidente. Già prima, nel 2008, le Nazioni Unite avevano considerato il Vajont come uno dei più grandi disastri causati dall'uomo, definendolo un «racconto ammonitore» con una parola, «evitabile», che brucia fortissimo. Ecco, penso che oggi dobbiamo ricordarci di tutto questo. Qualcosa del genere non deve più accadere. Dobbiamo mantenere viva la memoria di quel che accadde e delle responsabilità, anche con gesti concreti. Per esempio, il Governo con un proprio provvedimento deve stabilire che in modo definitivo il territorio bellunese diventi la sede degli archivi processuali. A sessant'anni dalla tragedia del Vajont, in una giornata in cui voglio credere che siamo tutti accomunati da uno stesso sentimento, valgano per noi quelle parole che scrisse proprio Tina Merlin: non si può soltanto piangere, è tempo di imparare qualcosa». la parola ricordo ha una etimologia molto importante nella nostra lingua: significa rimettersi nel cuore qualcosa, delle persone, delle comunità, dei momenti. La vicenda del Vajont ci interpella costantemente ed è una delle questioni che non possono essere derubricate, né tantomeno possono essere affidate all'oblio del tempo. Al contrario, per la sua drammaticità ma anche per la sua straordinaria contemporaneità, interpella l'uomo di oggi e la società di domani. È una ferita che rimarrà indelebile, certamente per le comunità di quelle montagne friulane e venete che vennero devastate dalla cupidigia e dalla voglia di risorse, di denaro, di successo, che poneva il tema del rispetto del territorio, della relazione con le comunità, del rispetto delle persone in secondo piano rispetto all'esigenza - come si direbbe oggi - di fare cassa. Ma è una ferita indelebile per l'intera comunità nazionale, perché la questione del dissesto idrogeologico, dello sviluppo sostenibile e dell'equilibrio tra la capacità di fare impresa e la tutela del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema, è oggi una sfida ancora più consistente, resa impellente dai cambiamenti climatici e dal grado di urbanizzazione che il nostro Paese ha raggiunto. Allora ricordare il Vajont, quelle comunità, quelle persone ad una ad una, perché ogni persona è preziosa, significa anche rimetterci nel cuore l'esigenza di dover costruire un'Italia di domani in cui non solo queste cose non avvengano più, ma in cui quelle esperienze siano uno straordinario monito affinché tutto ciò che si è verificato non si verifichi mai più. In questo senso e con questo spirito, ricordiamo il dramma di quelle comunità.

l'unico bellunese presente in Aula, non condividere le parole dei senatori Martella e Borghi quando parlano di una comunità profondamente ferita e lacerata da quello che è successo quella notte di sessant'anni fa. Per ogni bellunese, anche per quelli che come me nascevano qualche anno dopo, il Vajont segna una ferita che non si è ancora rimarginata; una ferita che tutte le generazioni del dopo-Vajont hanno curato e cercato di lenire. Hanno curato attraverso la memoria, attraverso i tanti comportamenti di

il tanto dolore, che non è solo il dolore di chi ha perso qualcuno in quella tragedia, ma è anche il dolore di chi ha visto poi scarse assunzioni di responsabilità in quello che è stato il *post* tragedia. Vi furono solo due condanne per la più grande tragedia ambientale italiana, dovuta

che toglieva ogni responsabilità all'uomo. No, lì l'uomo ebbe grandissime responsabilità, ed ebbe anche la grande responsabilità di non ascoltare i territori. Questo credo sia il primo monito che dobbiamo

dalle relazioni dei geologi, ma tanto anche dal sapere tramandato dalle generazioni. È per questo che ogni bellunese, quando si parla di acqua, quando si parla di dighe, quando si parla di invasi, si comporta come quella gatta che si è scottata con l'acqua calda, ma che oggi ha paura anche di quella fredda, perché questo è quello che si vive ancora a Belluno e vivono sulla pelle tanti bellunesi. due giorni fa si è recato proprio sulla diga, soprattutto in memoria delle persone che non ci sono più. Servono anche atti concreti come quello che citava prima il collega Martella riguardo agli archivi: non è una contrapposizione con chi oggi è all'archivio e che la legge dice essere il custode dell'archivio, cioè l'archivio di L'Aquila, che è stata la sede dei processi. È semplicemente

Signor Presidente, onorevoli senatori, sono trascorsi sessant'anni dal 9 ottobre al 1963, quando la nostra terra venne lacerata da una ferita tremenda che non si è mai rimarginata. Da quel giorno i nomi di Vajont, Erto, Casso, Longarone sono scritti nella storia del nostro Paese e sono entrati in maniera indelebile nei nostri cuori e nella memoria collettiva di tutti gli italiani. Sessant'anni fa la tragedia del Vajont ha spezzato la vita di 1.910 persone e ha cambiato per sempre la storia della nostra terra; una tragedia che è stata causata dalla colpevole presunzione degli uomini che volevano piegare la natura ai loro interessi economici. Lunedì, insieme al presidente Mattarella, ci siamo riuniti sul Vajont per ricordare le persone che non ci sono più, ma anche tutti coloro che sono rimasti e si sono rimboccati le maniche per ricostruire ciò che era stato distrutto. Rivolgo alle vittime un deferente ricordo e una preghiera. Rinnovo i nostri sentimenti di vicinanza alle loro famiglie e a tutti i sopravvissuti e dedico un pensiero di immensa gratitudine ai tanti soccorritori dell'epoca. È nostro dovere non dimenticare mai le vittime del Vajont e lottare perché disastri del genere non avvengano mai più.

in cui 1.910 cittadini veneti furono travolti e uccisi. Molte sono le riflessioni che si possono fare, colleghi, e in parte sono già state fatte dagli oratori che mi hanno preceduto. però vorrei porre all'attenzione un particolare secondo me estremamente significativo. La frana ebbe luogo nel monte Toc e già dal nome, che ha un carattere onomatopeico, si capisce la fragilità di quel territorio. quel nome non seppe interpretarlo, era un toponimo che risaliva alla cultura locale. In realtà, degli studi confermarono che quella è una terra molto fragile che non poteva sopportare un intervento come quello della diga, che peraltro era un manufatto pregevole dal punto di vista ingegneristico, tanto che sopravvisse alla tragedia. Chiunque risale la valle del Piave - penso che lo abbiamo fatto quasi tutti in quest'Aula - ad un certo punto, voltando lo sguardo a destra, non può che rimanere colpito da quella da quella diga, da quella grande opera ingegneristica che si staglia in quella direzione. Detto questo, io credo che noi non possiamo che trarre ammonimento da un evento così tragico. Prima di realizzare opere e interventi

ancor di più l'impresa eroica degli alpini, che anche in quell'occasione furono i primi soccorritori, furono fratelli delle vittime, si sporcarono nel fango e compirono un ulteriore gesto della loro grande epopea storica. *(Applausi)*.

Chiunque abbia fatto visita alla diga sa che l'ultimo pezzo della camminata per arrivare all'inizio del manufatto è costeggiato da uno steccato in legno che funge da parapetto e porta un filo su cui sono appesi dei foglietti di carta con i nomi dei bambini morti in quella tragedia. Quei nomi stanno lì a ricordarceli, ma credo abbiano una funzione più alta. Quella tragedia non è stata il frutto di sottovalutazioni, di un errore progettuale o di un'incapacità: è stata il frutto della cupidigia. Tutti conoscevano perfettamente i rischi di quell'intervento. E allora la domanda, oltre al ricordo che ci portano quei biglietti colorati con i nomi dei bambini, è soltanto una: saprà l'uomo fermarsi, qualche volta, di fronte a un rischio che porta però un grande beneficio economico? Se non saremo in grado di farlo, quel ricordo sarà un ricordo sprecato.

Avverto che per tale deliberazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea. Pertanto, la votazione della proposta di risoluzione avrà

96 della Costituzione, nei confronti del dottor Corrado Clini, nella sua qualità di Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore*. Invito i senatori Segretari a

sezione IV penale. Con il ricorso depositato il 7 febbraio 2023, il tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del senatore della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea nella seduta del 16 febbraio 2022 ha dichiarato l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 175 del 21 giugno 2023, depositata in cancelleria il successivo 27 luglio 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 14 settembre 2023. Nella seduta del 3 ottobre 2023 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso all'unanimità parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte Costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Sta a noi decidere se vogliamo che il Senato vada davanti alla Corte costituzionale a difendersi o se vogliamo che il procedimento prosegua con il Senato contumace. immunità parlamentari ha deliberato all'unanimità che il Senato si presenti, anche per rispetto, davanti alla Corte costituzionale a difendere le sue ragioni.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti. Poiché nessuno chiede di intervenire, con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Catania, sezione IV penale. *(Segue la votazione).*

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Presidente, l'azzardopatia è una piaga terribile che sta colpendo il nostro Paese, diventando ogni giorno sempre più grave. Gli ultimi dati fotografano una realtà molto preoccupante, con una crescita di fatturati altissima all'interno del nostro territorio.

136 miliardi drenati dalle famiglie più in difficoltà del nostro Paese: una cifra impressionante. Le persone che utilizzano questi soldi spesso e volentieri sono proprio quelle più in difficoltà, che dietro

Si parla in quest'anno di quasi di 80 miliardi giocati *online*. E lo Stato cosa fa? Lo Stato in realtà è biscazziere, perché dietro questa cifra trae profitto, quasi 10,3 miliardi di euro presi da queste persone molto in difficoltà. E sta quasi chiudendo gli occhi di fronte a quelle *lobby* che in questo momento spennano i nostri cittadini. Questi sono i dati ufficiali. I dati più preoccupanti sono quelli che non sappiamo e che non vediamo, sono quelli difficili da calcolare, cioè sono proprio quelli del bilancio sociale. Non sappiamo qual è il costo sanitario che c'è dietro a tutto questo: quante famiglie distrutte, quante persone, quanti giovani dietro il gioco *online* stanno cadendo in questa piaga sociale? Abbiamo la responsabilità, in questa fase, di intervenire, di affrontare e di impedire che una cifra del genere finisca dentro un'industria che non porta a nulla e che sottratta a famiglie che sono estremamente in difficoltà. Termino, Presidente, dicendo che misureremo la volontà di questo Governo con atti emendativi, per vedere se sono dalla parte dei cittadini o dalla parte delle *lobby*. Lo stiamo vedendo tutti i giorni come stanno cercando di aggirare le leggi che sono state fatte durante il Conte I. Come stanno cercando di aggirare le leggi lo vediamo in ogni partita di calcio, in ogni gioco pubblico alla televisione, dove stanno eludendo le leggi che abbiamo fatto. Quindi sul decreto Caivano inseriremo dei testi che andranno a impedire questo aggiro delle norme. *(Applausi)*.

è passato a nuova vita il senatore Francesco Salzano, una persona perbene, che ha rappresentato veramente il popolo in quest'Aula, nella XIV legislatura. Un medico che ha onorato veramente il suo giuramento ad Ippocrate, perché era sempre pronto

Francesco Salzano è stato anche un autorevole esponente politico, punto di riferimento per la sua città, Nocera Inferiore, dove è stato per svariati anni

legislatura, compiendo un'impresa, perché, da candidato del partito Democrazia Europea, riuscì ad entrare in Senato in quella lista che non vide eletto neanche il segretario nazionale. Questo a dimostrazione di un consenso personale straordinario, che fu notizia in Italia. Il senatore Salzano è stato veramente una persona di grande equilibrio, mai un equilibrista, moderato per costituzione morale e politica. È stato una persona animata da un sincero senso civico e spirito di servizio. Ricordo lo *slogan* di una sua campagna elettorale, che recitava: è colpevole chi può fare e non lo fa. Quella frase dipinge perfettamente l'uomo e il politico. Egli lascia, in tutti noi che lo abbiamo conosciuto, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerlo, un grande vuoto di vita. Pertanto, vorrei rivolgere alla sua amata famiglia, alla moglie, ai figli, al fratello, ai nipoti, il più sincero abbraccio, e dire che non mancherà soltanto a loro l'uomo, Francesco, ma mancherà anche a noi il medico e il senatore della Repubblica, Salzano. *(Applausi)*.